Onorevoli colleghi, il senatore Sergio Vetrella, con lettera pervenuta in data 13 luglio 2010, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di senatore, optando per la carica di assessore della Giunta regionale campana. Trattandosi di un caso di opzione derivante da una situazione di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, il Senato non può che prenderne atto. Per consentire alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di procedere agli accertamenti relativi all'individuazione del candidato subentrante, autorizzo la stessa Giunta a convocarsi sin d'ora.

nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Tancredi. Ne ha facoltà. Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, dopo un lungo, laborioso e proficuo lavoro della Commissione bilancio, la manovra correttiva di finanza pubblica di cui stiamo discutendo approda in quest'Aula. Con soddisfazione vorrei preliminarmente sottolineare che, proprio poche ore fa, l'Italia ha ricevuto il riconoscimento da parte dei Ministri dell'ECOFIN dell'adeguatezza dei provvedimenti finora adottati: in altre parole, l'Unione ha dato al nostro Governo di aver preso misure effettive ed adeguate, perfettamente in linea con gli impegni assunti, in coerenza con quel Patto di stabilità e di crescita che costituisce presupposto necessario per 1'esistenza stessa dell'Europa. La ragione della politica di rigore, cui la manovra si ispira, trova quindi conferma nella menzione positiva ricevuta dall'Unione europea e dai mercati. Si tratta di una conferma importantissima, visto che si è parlato in questi giorni di finanziaria europea e che tutti hanno enfatizzato l'importanza dell'organicità di questo provvedimento all'interno della politica comunitaria. Deve essere dunque impegno di tutti tutti dare al Paese prova di serietà e di responsabilità, penetrare nella coscienza dei cittadini e trasmettere loro che il doloroso programma di austerità è non solo il prezzo della partecipazione all'Eurozona, ma la garanzia più sicura della stabilità a lungo termine, la necessaria tutela del nostro sistema strutturale, l'unica strada percorribile per assicurare la sostenibilità della finanza pubblica. Questa manovra non è la tradizionale operazione di aggiustamento dei conti pubblici, ma costituisce una riduzione del peso dello Stato nell'economia e nella società: una riduzione necessaria in un'ottica liberale, per tagliare costi e sprechi e per reperire maggiori risorse da destinare alla crescita ed alla creazione di un sistema Paese competitivo, con meno burocrazia e più efficienti misure di stimolo alla ripresa economica. Dal lato della spesa, gli aggiustamenti si sostanziano essenzialmente in una rilevante riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione, oltre all'inevitabile sacrificio richiesto ai dipendenti pubblici, quale necessario bilanciamento di una posizione comunque privilegiata rispetto ai lavoratori privati. un atto di responsabilità doveroso per tutti coloro che godono della certezza di un posto di lavoro, che non scontano gli squilibri del mercato con licenziamenti e cassa integrazione e che, in quanto dipendenti dello Stato, devono con coscienza e serietà partecipare al suo risanamento. Si è chiesto anche alle Regioni, alle Province ed ai Comuni di ridurre le spese meno produttive, ai Ministeri di rimodulare le risorse destinate alle proprie strutture, agli apparati politici e amministrativi, in buona sostanza, il contenimento e la razionalizzazione dei *budget* di loro pertinenza. Per dirla con Croce, si è dovuto combattere «taluni eccessi di socialità burocratica e spendacciona», controllando con più rigore la spesa pubblica, al fine di rendere operativi quei criteri di razionalità e di efficienza a favore dei bisogni sociali più immediati e concreti. Voglio sottolineare che al rilancio ed alla ripresa economica è orientata la nostra manovra, che non trascura la valorizzazione dell'iniziativa privata e della libertà di impresa, riconoscendo in tali valori la propulsione irrinunciabile di ogni virtuosa economia. È questo il senso della SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività, che sostituirà gran parte dei regimi di autorizzazione rinviando i controlli amministrativi ad una fase *ex post*. Ed è questa altresì la *ratio* sottesa alla possibilità riconosciuta alle imprese di compensare i crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione con Dal lato delle entrate, invece, la manovra è stata principalmente concepita sulla base del potenziamento dei processi di accertamento e riscossione dei tributi e delle misure antievasione. Il contrasto all'attività evasiva è un obiettivo da perseguire sul piano dell'efficienza economica, oltre che su quelli dell'equità e della legalità. Non può, tuttavia, non rilevarsi che l'instabilità economica, nell'evoluzione delle economie europee, è ormai un fenomeno fisiologico; sulla complessità strutturale della scena economica agiscono nuovi e vecchi attori, che non possono interpretarsi con categorie e stereotipi precostituiti. Occorre allora riflettere criticamente sui cambiamenti della struttura produttiva del sistema, evitando di innescare pericolosi meccanismi che mettano a rischio la crescita, inadeguati a fornire una risposta a fenomeni, processi e mutamenti globali, non all'altezza dei tempi che stiamo vivendo. Per concludere, vorrei ribadire la necessità di un nostro impegno, di un impegno della politica e delle istituzioni verso lo sviluppo di riforme strutturali, orientate sì a ridurre il *deficit*, ma attente, al contempo, a non danneggiare lo sviluppo e l'occupazione. Diamo concretezza a quei *global legal standard* che 34 Paesi aderenti all'OCSE hanno recentemente approvato, principi di etica, trasparenza e correttezza di cui i mercati e la finanza mondiale non possono ormai più fare a meno. Ritroviamo il cammino della crescita su un terreno condiviso, in cui poche, ma chiare regole etiche e legali, che auspico poter essere trasfuse in un trattato internazionale multilaterale, siano l'antidoto contro il ripetersi di crisi sistemiche e la garanzia di una maggiore solidità ed equità dei mercati. Mi è d'obbligo dedicare gli ultimi minuti del mio intervento alla questione del terremoto in Abruzzo. La norma perfezionata dalla Commissione, contenuta nell'articolo 39, è solo l'ultimo passo di un cammino ancora lungo di provvedimenti messi in campo dal Governo fin dalle prime ore successive al terribile sisma del 6 aprile 2009. Inizialmente, si sono investite tutte le risorse per assicurare a tutti i cittadini dell'Aquila una dimora stabile, nel più breve tempo possibile, operazione riuscita brillantemente e che è oggettivamente difficile contestare. Nello stesso tempo, si è fatto in modo che, a settembre, tutte le scuole aquilane e del cratere potessero ripartire, obiettivo anche questo raggiunto brillantemente. Altra misura importante è quella di aver assicurato a tutti i lavoratori dipendenti un reddito, con un massiccio ricorso agli ammortizzatori in deroga; ma anche per i lavoratori autonomi è stato previsto ed erogato un sussidio fino a quando non avessero riattivato le proprie attività. Come in altre situazioni simili, c'è stata la sospensione delle tasse e dei contributi previdenziali per tutti i cittadini e le imprese del cratere, sospensione che si è protratta fino al 30 giugno scorso. L'articolo 39 della manovra rinvia l'inizio della restituzione delle tasse e contributi non pagati al 1° gennaio 2011 e prolunga la sospensione a dicembre 2010 solo per i lavoratori autonomi e per le imprese con volume d'affari al di sotto dei 200.000 euro. Riguardo alla dilazione della restituzione ed anche ad un eventuale sconto sulle somme da restituire, c'è un impegno di autorevolissimi esponenti del Governo ad intervenire con norme specifiche, in questo ed in futuri provvedimenti legislativi, da porre in essere comunque prima del 1° gennaio 2011. Le risorse impegnate per far fronte a tali misure sono ingenti (617 milioni di euro) e assorbono integralmente le entrate dovute alla seconda fase dello scudo fiscale. A mio modo di vedere, non costituisce una priorità l'ulteriore sospensione dei pagamenti fiscali e contributivi per i lavoratori dipendenti - so che su questo argomento sono abbastanza isolato ma la penso così - visti anche i dati del Ministero dell'economia che evidenziano sul territorio aquilano un aumento dei depositi bancari nell'ultimo anno. Le problematiche che il Governo si trova ad affrontare in questo momento sono invece complesse e di difficile soluzione; si tratta di avviare a pieno regime la ricostruzione e di aiutare la ripresa del tessuto economico aquilano. Il ripristino della zona franca ed il raddoppio della sua dotazione finanziaria (da 45 a 90 milioni di euro), anch'esso contenuto nell'articolo 39 - e introdotto con un emendamento *bipartisan* che dovrebbe essere ad esempio dell'azione politica da mettere in campo su questa difficile materia - danno sicuramente una prima importante risposta alla seconda esigenza. Per quanto riguarda la prima, la ricostruzione, cioè, non esistono, in realtà, problemi di disponibilità di risorse. La ricostruzione può essere finanziata con il fondo di 2 miliardi di euro messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti, ad anticipo del fondo, di cui all'articolo 14 del decreto Abruzzo. Prova ne sono i pochi significativi interventi privati, già partiti e finanziati, anche se pochi. Mi risulta che molte istruttorie si stanno compiendo anche su edifici di tipo E, i più danneggiati. Esiste sicuramente un problema, non banale, di *governance* da parte del Comune dell'Aquila e degli altri Comuni del cratere, certamente impreparati, nelle loro strutture, a gestire una problematica così complessa. Ritengo che, in maniera sussidiaria, il Governo, anche attraverso la struttura di missione del commissario delegato, debba essere messo in condizione di assistere e coadiuvare gli enti locali. La ricostruzione di un tessuto urbano, così profondamente ferito come quello aquilano, non è esercizio banale e siamo tutti consapevoli che richiederà del tempo. È sulla via della soluzione, in questi giorni, un'altra criticità evidenziatasi negli scorsi mesi: la carenza di risorse a disposizione del commissario delegato per onorare gli impegni presi dalla gestione dell'emergenza (puntellamenti, interventi d'urgenza, contributi di autonoma sistemazione). Il Ministero dell'economia ha garantito lo sblocco di diverse centinaia di milioni di euro, sufficienti a soddisfare le tante imprese che si trovano scoperte da qualche mese, avendo anticipato lavori e servizi. In esito a questa sintesi, ritengo che la classe politica aquilana, abruzzese e dell'intero Paese, debba impegnarsi in maniera seria nella ricerca di soluzioni utili alla rinascita dell'Aquila. Credo che isterismi, voglia di visibilità di questo o quel personaggio politico, di destra o di sinistra, verificatasi nelle ultime settimane, non contribuiscano a risolvere la situazione, ma anzi aumentino le ansie e le paure di una popolazione così gravemente colpita. pur consapevole delle inefficienze inevitabili verificatesi in questi 15 mesi e dei gravi disagi che ancora oggi deve sopportare la popolazione aquilana, penso che il Governo e la maggioranza debbano essere orgogliosi del lavoro svolto fino ad oggi, forse senza precedenti nella gestione di emergenze simili.

colleghi, rappresentanti del Governo, la situazione dei conti pubblici è critica ed era necessaria una manovra correttiva.

miliardi; un *deficit* superiore al 5 per cento, una crescita molto bassa, appena sopra di qualche decimale dello 0,5 per cento; una disoccupazione che cresce, e che colpisce soprattutto i giovani e le donne;

Il nostro Paese tiene dal punto di vista economico e finanziario perché gli italiani sono delle formichine. A causa del risparmio privato, l'indebitamento delle famiglie è molto più basso rispetto a quello degli altri Paesi occidentali: questa è la situazione e la realtà.

Questa manovra aiuta la crescita? Assolutamente no, in quanto deprime la crescita, è una manovra regressiva.

corressero in parallelo in modo che quando si arriverà a discutere di federalismo fiscale effettivamente si realizzino i presupposti e gli agganci per poterlo fare bene. La manovra incentiva gli investimenti? Assolutamente no.

significativo alla ripartenza del volano del settore edilizio o del settore delle costruzioni. La manovra corregge l'anomalo funzionamento dei pagamenti nella pubblica amministrazione? Assolutamente no. Noi accettiamo che la pubblica amministrazione paghi di più beni e servizi perché è sottinteso che essa paghi a distanza di sei mesi o addirittura di un anno. È un'assoluta incongruenza rispetto all'obiettivo che

assumono; una tassazione più severa nei conferiti delle rendite finanziarie, perché di fatto questo Paese è solo ed unicamente sulle spalle dei lavoratori dipendenti e delle persone a reddito fisso; una riduzione della spesa corrente che non sia fatta in termini lineari ma che vada realmente ad incidere sugli sprechi. Per fare questo dobbiamo fare un'analisi, capitolo per capitolo, di ogni bilancio, settore per settore, servizio per servizio di ogni Ministero, di ogni Regione e Comune per far questo serve un Patto di stabilità che responsabilizzi sindaci, funzionari, dirigenti, non meccanismi lineari che non danno alcun tipo di responsabilità. Infine, voglio soffermarmi sulla questione relativa agli enti locali e territoriali.

gli enti territoriali come un peso per questo Paese? All'interno della pubblica amministrazione, siete veramente convinti che di tutto il comparto la parte peggiore sia quella costituita dagli enti territoriali, quindi la periferia?

e quel che abbiamo chiesto è un patto di stabilità completamente diverso, più responsabile. Viceversa, se continuate in questo modo l'anno prossimo si porrà in essere una vera e propria macelleria sociale all'esterno,

intervengo anch'io sul contenuto della manovra che il Governo porta all'esame del Parlamento non senza omettere di far rilevare che la manovra si rende necessaria in una condizione di depressione economica a livello internazionale e mondiale, con un calo del prodotto interno lordo del nostro Paese che finora però non aveva portato ad una decurtazione delle spese, in particolare della spesa pubblica.

per esempio, un aumento della presenza italiana nel commercio internazionale. La quota italiana è salita a 4,9 per cento, subito dopo la Germania: c'è da augurarsi che la ripresa economica stia anche nel nostro Paese coinvolgendo i settori manifatturieri più importanti e che riguardano le esportazioni. Tuttavia, nel dibattito che si è svolto in Parlamento è emerso uno spaccato molto critico nei riguardi della manovra operata dal Governo e, in particolare, sul settore del del pubblico impiego e della pubblica amministrazione. Anche nella mia qualità di sindaco, io ritengo che la manovra dovesse tener conto in modo più puntuale delle esigenze degli enti locali. Ciò nondimeno, i i Comuni più virtuosi, quelli che hanno rispettato il Patto di stabilità, potranno conseguire quelle economie, anche interne, e quella razionalizzazione della spesa che potrà far sì che i Comuni eroghino quei servizi indispensabili ai cittadini che la nostra Costituzione prevede, secondo il principio di sussidiarietà verticale, siano di stretta competenza degli enti locali.

Per quanto riguarda più segnatamente gli interventi relativi al comparto della sicurezza (e in questa sede molti colleghi si sono spesi a difenderne gli interessi),

530 milioni per finanziare la legge sui parametri e la restante parte per riconoscere il principio di specificità del settore rispetto al pubblico impiego. principio di specificità è norma che, con un provvedimento collegato alla finanziaria, questo Governo sta portando all'approvazione del Parlamento. Ciò nondimeno, non vorrei si dimenticasse che, nel breve periodo in cui il Governo del centrosinistra governò l'Italia, nel 2007

Sempre segnatamente al personale del comparto sicurezza e difesa, vorrei ricordare che la manovra lascia inalterato il *plafond* complessivo

cerca di finanziare il mancato incremento retributivo derivante dalle promozioni in carriera di questo personale.

ma, per la prima volta, nonostante la crisi economica internazionale che ha portato la Grecia a tagliare una gran parte dei salari del personale pubblico, il Regno Unito a ventilare la possibilità di licenziare decine di migliaia

del disagio di quel personale. Pertanto, se le condizioni finanziarie ed economiche del nostro Paese miglioreranno, si potrà operare una revisione successiva con le prossime leggi finanziarie. Non sono abituato a fare demagogia. Nella mia esperienza, anche professionale, di rappresentanza ultraventennale so che mai questo settore ha conosciuto momenti di vacche grasse. Abbiamo sempre fatto una contrattazione collettiva, tenendo conto delle risorse finanziarie, e non pochi sono stati i momenti gravi, come quelli che negli anni '90 portarono al governo del Paese

senatore Azzollini, relatore di tale complesso testo. In verità, stiamo conducendo un dibattito su un testo diverso da quello sul quale

perché mi riferisco - chissà - ad una speranza, molto recondita: ossia, che ancora sopravvivano nel maxiemendamento ipotesi testuali su cui tanto si è discusso

alcuna possibilità di recupero, della cultura, alla cultura, della comunicazione, alla comunicazione. La riduzione di trasferimenti alle Regioni, presidente Azzollini, è pari a 4 miliardi di euro per il 2011 e a 4,5 miliardi per gli anni successivi;

50 milioni di euro all'anno è il taglio per il Ministero dei beni culturali in attività che riguardano la tutela e la valorizzazione, quindi l'Italia, che è fatta in gran parte di beni culturali. Ho aggiunto tali dati a quelli che più frequentemente riportiamo, che comunque qui ripeto: il taglio del 50 per cento del finanziamento dei 232 enti culturali (quelli nelle tabelle), grandi e straordinari o meno grandi, ma non meno straordinari e importanti; il taglio secco, senza alcuna *pietas*,

Azzollini, sa essere circa quello che costa una cena tra amici per voi, che in genere andate in ristoranti di una certa quotazione. Dunque, l'Ente teatrale italiano, il teatro pubblico italiano, che assomiglia e fa quello che fanno tanti altri consimili in altri Paesi, è tagliato.

Signora Presidente, il mio contributo al dibattito sulla manovra intende sviluppare tre riflessioni. In primo luogo, la crisi globale che sta mettendo a dura prova i Paesi d'Europa; in secondo luogo, come sta reagendo l'Italia a questa crisi luogo, cos'altro si dovrebbe fare per consentire al Paese di coniugare la doverosa politica di rigore sui conti con la necessità di rilanciare lo sviluppo economico recuperando competitività. Per quanto riguarda l'origine della crisi, ho ascoltato molte opinioni; la mia valutazione è che la crisi globale nasce dalla più grande bolla immobiliare finanziaria degli ultimi decenni, che è stata alimentata da un'autentica esplosione dei debiti privati. Secondo fonti autorevoli, tra il 2000 e il 2008 la crescita del debito aggregato pubblico e privato nelle principali economie avanzate è stata di oltre 40.000 miliardi di dollari; il 75 per cento di tale aumento è stato generato non

nel 2007 con lo scoppio della bolla immobiliare e finanziaria ed il conseguente fallimento del più evoluto sistema finanziario del mondo, quello americano; nel 2008 la crisi da finanziaria diventa crisi dell'economia reale e, nel maggio

finanziaria, dando prova di avere un sistema bancario che ha retto sul campo; essa ha infatti dimostrato una grande solidità, se è vero, come è vero, che le banche italiane hanno resistito allo tsunami del 2008 senza ricorrere ad aiuti dello Stato. C'è stato - è vero - un atteggiamento positivo del Governo, che ha funzionato molto bene quando è stata data assicurazione che mai un risparmiatore avrebbe rimesso un euro dei propri risparmi depositati nelle banche italiane. Il Governo statunitense ha dovuto invece indebitarsi per proteggere, tutelare, difendere le proprie banche, mettendo a disposizione oltre 2.000 miliardi di dollari; il Governo inglese ha stanziato poco più di 500 miliardi di sterline per salvare il proprio sistema bancario, arrivando, ahimè, a nazionalizzare sei grandi banche inglesi. La trincea dura della crisi ha quindi reso giustizia al sistema bancario italiano, tante volte ingiustamente

prestigiosi editorialisti di quei giornali sparavano sulle banche italiane, accusandole di non saper parlare inglese, di non aver cioè seguito - e, *a posteriori*, dico «per fortuna» - il modello anglosassone nel fare banca. Le banche italiane, quindi, con la regia autorevole della Banca d'Italia, non hanno obbedito a questi richiami e hanno superato indenni la bufera. Per quanto riguarda la crisi dell'economia reale, la crisi finanziaria, con la stretta creditizia conseguente, ha generato nel 2009 la crisi dell'economia reale; si è avuto un crollo del commercio mondiale, un crollo del PIL ed un aumento considerevole della disoccupazione.

della triennalità della manovra. La manovra si è qualificata soprattutto per uno stanziamento cospicuo a favore della cassa integrazione guadagni di 7 miliardi di euro per l'anno 2009. Si è così allargato l'ombrello della protezione sociale verso quei lavoratori esclusi dal sistema produttivo

non si sono avute nuove manifestazioni di protesta, non si sono svolte occupazioni di fabbrica, insomma, c'è stata una gestione politica della crisi economica che ha badato soprattutto a privilegiare la cosiddetta coesione sociale.

e cominciavano ad apparire i primi barlumi di una luce in fondo al tunnel, quasi a voler significare che stavamo uscendo dalla crisi dell'economia reale, è scoppiato il finimondo nella prima settimana, in particolare nei giorni 8 e 9 maggio: i giorni terribili dell'attacco della speculazione internazionale all'euro e all'Europa.

quindi una condizione particolare per cui, a fronte di istituzioni che reggono, non esiste una politica convergente da parte di tutti i Paesi componenti l'Unione europea. delle rispettive politiche di bilancio, delle rispettive politiche fiscali, della spesa pubblica, sia nazionale che locale, degli incentivi, delle retribuzioni, dell'organizzazione del *welfare.* Insomma, l'Europa si dimostra, purtroppo, ancora lontana dall'esserci data una struttura federale e politiche comuni

Quindi, i mercati, la speculazione internazionale, hanno segnalato con forza che tale prospettiva è insostenibile. Come dice Tremonti, è per questo che ci troviamo di fronte ad un tornante della storia. Non possiamo continuare a vivere come se nulla fosse. Per questo i 24 Paesi dell'Unione europea

coloro che accusano il Governo italiano di non aver saputo prevedere la crisi finanziaria peccano di cecità. Nessuno ha saputo prevedere quello che sta accadendo in questi giorni, in queste settimane.

dobbiamo prendere atto che la crisi ha una dimensione internazionale e che dalla crisi si esce non solo e non tanto con risposte e decisioni del Governo nazionale, ma soprattutto con decisioni che devono essere prese a livello europeo. Ha fatto bene il Governo, all'unisono con gli altri Paesi europei, ad avviare scelte e decisioni rigorose e impopolari, sottoposte all'attenzione del nostro Paese e di questa Assemblea, come ben hanno ricordato sia il relatore di maggioranza che il relatore di minoranza, e la cosa non è priva di significato. Ci sono quattro punti nei confronti dei quali c'è condivisione - anche in quest'Aula, ritengo - tra maggioranza e minoranza: la necessità e l'urgenza di questa manovra correttiva, il riconoscimento

Certo, manca il tempo tecnico e manca a me in questo momento il tempo per sviluppare ulteriori riflessioni. Mi avvio alla conclusione, signora Presidente, però devo dire una cosa. Io non credo che una manovra fatta di soli tagli di contenimento della spesa possa essere considerata necessaria e sufficiente. Sicuramente è necessaria, ma non è sufficiente. Per questo mi sono battuto in Commissione per introdurre modifiche normative che fossero finalizzate alla ripresa dello sviluppo, che fossero finalizzate a far sì che venissero riavviate politiche di investimento, soprattutto in tre settori strategici: i porti, gli aeroporti e le opere pubbliche. Io credo che occorra riprendere con forza la via delle riforme strutturali in quei settori vitali del nostro sistema produttivo; quelle riforme che recentemente ci ha ricordato il Governatore della Banca d'Italia. Occorre soprattutto, signora Presidente, fare con convinzione un salto culturale nel campo delle opere pubbliche. Se non possiamo più contare su risorse aggiuntive per sostenere una politica di ripresa degli investimenti, allora dobbiamo creare le condizioni legislative in forza delle quali le infrastrutture in grado di generare reddito debbano essere in Italia progettate, costruite e gestite da operatori privati, ai quali va detto che il ritorno dell'investimento lo avranno garantito proprio con la gestione delle infrastrutture stesse. Dopo la positiva esperienza della legge n. 166 del 2002 che ha introdotto dopo il terzo correttivo del 2008, noi possiamo dotarci di un corredo normativo ancora più avanzato. Dopo i 10 miliardi che i privati hanno investito nel 2009 e i 25 miliardi che sono stati investiti in opere pubbliche dai privati dal 2003 al 2008, possiamo immaginare

che questa manovra, doverosa e necessaria, non è sufficiente per rimettere il Paese in grado di competere nella sfida dell'economia globale. Dobbiamo smetterla di riconoscere il nostro Paese come il Paese del debito pubblico. L'Italia è certo un Paese che ha un debito pubblico significativo, ma è anche il Paese che ha la più grande quantità di risparmio privato accumulato, il più solido e robusto sistema finanziario e bancario d'Europa e il maggior numero di imprenditori che non chiedono altro se non la capacità di investire, avendo regole precise, procedure certe e tempi di realizzazione sicuri.

prospettive di sviluppo e futuro al Paese. Ha colpito la scuola, l'università, la ricerca, che sono la chiave di volta per uno sviluppo economico di qualità, per l'occupazione, per la coesione sociale, per i diritti e le pari opportunità delle persone. Non è intervenuto per sostenere l'occupazione dei giovani e delle donne, che sono un patrimonio essenziale di risorse innovative e creative. Ha tagliato i servizi essenziali, non le strutture burocratiche. Basti pensare che non è stato accolto l'emendamento del Partito Democratico che proponeva il raggruppamento degli uffici periferici dello Stato La manovra colpisce gli enti locali e i sistemi territoriali, che sono l'ambito territoriale e la leva per lo sviluppo locale, per la valorizzazione delle inestimabili risorse ambientali, creative, culturali, economiche del nostro Paese. È una manovra inadeguata e debole, ed insieme è una manovra ingiusta, perché esclude dai sacrifici chi ha di più. Esclude le rendite finanziarie e i grandi patrimoni e colpisce chi ha di meno, i più deboli. Perché, ad esempio, non è stato accettato un emendamento, da noi proposto, che prevedeva di stabilire un prelievo di solidarietà triennale del 5 per cento su tutti i redditi superiori ai 150.000 euro? Sarebbe stata un'entrata che avrebbe coperto e sostituito tanti dei tagli che invece vengono fatti. Voglio esemplificare come si colpiscono i più deboli, con due esempi in particolare. disabili, è vero che l'emendamento del relatore ha cambiato la percentuale delle invalidità per le pensioni e l'assegno di accompagnamento; ma rimangono, e anzi sono state aggiunte, norme pesantissime contro l'integrazione scolastica degli alunni disabili. Ne cito tre: il tetto per il numero complessivo degli insegnanti di sostegno, fissato per legge e già dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte sono state irrigidite le norme per le commissioni che devono certificare l'invalidità e la non autosufficienza dei ragazzi per l'attribuzione degli insegnanti di sostegno; da ultimo, con un emendamento viene annullato il limite massimo di 20 alunni quando nella classe c'è un ragazzo disabile. Lette insieme, queste tre norme individuano un vero accanimento del Governo nei confronti dei più deboli tra i deboli: i bambini e i ragazzi disabili, che hanno il diritto di imparare e crescere insieme con i loro coetanei. È la buona integrazione scolastica, un vanto per il nostro Paese, che viene concretamente messa in discussione; così il Governo apre la strada a percorsi separati e segreganti. Secondo esempio: la manovra grava in modo ingiusto e inaccettabilmente pesante nei confronti del personale della scuola; infatti, sono solo i docenti e il nel pubblico impiego che è stato particolarmente colpito da questa manovra, a subire danni permanenti sugli stipendi, sulle pensioni e sulla liquidazione.

320 milioni di euro soltanto il primo anno, 640 il secondo, 960 il terzo, un miliardo 920 milioni di euro, oltre 18 miliardi di euro calcolati finché la manovra avrà effetti, cioè fino al 2047. È possibile che questo accada nel silenzio generale? Un emendamento del relatore stabilisce inoltre che attraverso un decreto interministeriale si definirà l'utilizzo,

miliardi di euro che io auspico siano destinati a questo scopo, ma l'emendamento non lo dice e parla solo di un decreto interministeriale. Chiedo quindi al Governo qui

ma se il Governo avesse veramente avuto a cuore l'economia italiana, con tutta probabilità non si sarebbe comportato in maniera così autoritaria e non avrebbe eretto un muro di fronte alle istanze presentate non solo dall'opposizione, ma anche dalla stessa società civile, la quale

Non si capisce, dunque, la ragione per la quale il Governo abbia deciso di inserire questo disegno di legge nella manovra, né quale sia l'urgenza. Di nuovo, dunque, contesto il modo di agire della maggioranza che reputo assolutamente irrispettoso delle prerogative parlamentari riconosciute dalla Carta costituzionale. L'emendamento 4.1000, già approvato in Commissione bilancio, inserito in una manovra che applica tagli severi a settori strategici per il nostro Paese, prevede, paradossalmente, uno stanziamento di quasi 21 milioni di euro

era quella di diffondere i valori e la cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni. Mi chiedo e domando anche a voi, onorevoli si possa pretendere di trasmettere il valore intrinseco delle nostre Forze armate e della Patria in sole tre settimane, per di più attraverso dei corsi puramente pratici e fisici. Se malauguratamente così non fosse, allora, dovremmo seriamente preoccuparci per lo stato della difesa e per le sorti future del nostro Paese. Leggendo l'articolato, largamente ripreso dall'emendamento in questione, vengono i brividi e immediatamente torna alla mente quella famosa legge Balilla che il regime fascista approvò nel lontano 1926. Questo emendamento è persino peggiorativo di quella legge. I requisiti psico-fisici richiesti ai futuri partecipanti, infatti, sono di gran lunga più severi e selettivi di quelli che allora si chiedevano alle giovani leve. Al fine di poter frequentare questi corsi, infatti, un ragazzo deve, secondo quanto previsto dai Ministri in questione, essere idoneo all'attività sportiva agonistica. È un errore ed una vergogna, colleghi, sostenere che la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale non possa avvenire anche tra i giovani che, per motivi di salute o disabilità fisica, sono impossibilitati a svolgere attività sportive agonistiche. I valori legati alla Patria e alla pace non si trasmettono attraverso flessioni o esercitazioni fisiche. Per questo motivo noi dell' Italia dei Valori avevamo chiesto in Commissione che nell'arco delle tre settimane non fosse consentito l'uso delle armi e venisse, piuttosto, coinvolto il mondo accademico e costituzionalista. Ma le nostre istanze sono, purtroppo, rimaste puntualmente inevase, a conferma dell'intenzione puramente militaristica che ha mosso gli ideatori dell'emendamento. Vorrei portare alla vostra attenzione anche un altro aspetto. L'Esercito, come tutti voi saprete, è composto anche da volontari in ferma breve e in ferma prefissata. Un numero assolutamente rilevante di questi giovani ha prestato servizio nelle missioni internazionali tenendo alto il nome del nostro Paese. Al rientro in Patria però, dopo 4 o 5 anni di attività, molti di questi si sono accorti di aver sacrificato anni importanti della loro vita per una formazione che non servirà loro. Non vengono confermati e, a causa dell'assenza di fondi che possano permettere la loro stabilizzazione, vivono in uno stato di totale abbandono da parte dello Stato e vengono quindi rimandati a casa.

di questi giovani. In un momento poi in cui la crisi economica globale si fa sentire con la sua massima efferatezza, la razionalizzazione della spesa pubblica diviene ancora più difficile da compiere, ma strategicamente fondamentale per il Paese. Occorre capire dove sono le priorità e dove i vezzi. Bene, colleghi, io questo provvedimento lo definisco un capriccio, una macchietta ideologica che questo Governo ha deciso di compiere, per non dire una marchetta ideologico-fascista. Mi rammarico con il ministro La Russa per la poca autorevolezza che ha dimostrato in merito alla stesura di questo provvedimento. In maniera prona ha accettato tutti i tagli che a mò di accetta si sono abbattuti sul comparto sicurezza:

Sono tagli che non vanno ad incidere su un sistema funzionate ed ottimale perché, purtroppo, le condizioni nelle quali operano le nostre Forze armate sono già critiche. sono più, infatti, i fondi per finanziare l'addestramento e la formazione delle Forze armate, già tagliati del 40 per cento dal famigerato decreto-legge n. 112 del 2008. Gli agenti e i militari hanno ormai a disposizione pochi mezzi, spesso privi di pezzi di ricambio e persino di carburante. Si tratta dunque di scelte finanziarie dunque scellerate, come anche la mancata soppressione della società Difesa servizi spa, ulteriore centro di spesa che va a togliere finanziamenti vitali a comparti fondamentali che si trovano in situazioni di grave deficit, peraltro approvato con modalità analoghe a questa bella norma Balilla. Colleghi, lancio questo accorato appello: accantonate questo emendamento che ci riporta al periodo dei giovani Balilla, scindetelo dalla manovra. Date prova di essere almeno un po' responsabili di fronte alla gestione delle risorse pubbliche; date prova di avere quella sensibilità che fino ad ora non è emersa. Se i ministri La Russa, Tremonti e Meloni hanno a cuore l'istituzionalizzazione di questi corsi, allora chiedo loro di rispettare le prerogative parlamentari e lasciar proseguire l'*iter*, già iniziato in Commissione, di questo disegno di legge.

come e quanto il testo della manovra correttiva, approvato in Commissione bilancio, sia stato integrato e modificato. Nella sola seduta pomeridiana di venerdì scorso, sono stati esaminati numerosi emendamenti che erano stati accantonati in precedenti sedute. Verrebbe da pensare, vista la natura del provvedimento in discussione, che si sia trattato di proposte migliorative sulla lotta all'evasione fiscale, sui tagli alla spesa pubblica o, ancora, sulla soppressione di qualche Nulla di tutto questo: un intero pomeriggio di discussione e di votazioni è stato dedicato all'approvazione di emendamenti che vanno dalla soppressione dell'interpretazione autentica per chiarire le disposizioni sui benefici in favore dei soggetti colpiti dall'alluvione del '94 in Piemonte, alle disposizioni che prevedono che la prova di ammissione ai corsi universitari svolti in lingua straniera sia predisposta direttamente nella lingua medesima, alla previsione di modifiche del bando per la realizzazione dell'autostrada del Brennero, all'estensione della cassa integrazione nel settore della pesca. Tutti degnissimi provvedimenti, a ben vedere, ma - non per citare autorevoli uomini politici dell'altro ramo del Parlamento - qualcuno sa spiegarmi che «ci azzeccano» con una manovra correttiva che dovrebbe occuparsi essenzialmente di contenimento della spesa pubblica, lotta all'evasione fiscale e che eventualmente dovrebbe rimodulare la fiscalità in direzione di una maggiore equità? *Dulcis in fundo*, o *in cauda venenum* (scegliete voi): quando ormai la Commissione era giunta quasi alla fine del suo lavoro, sono comparsi tre corposi emendamenti (il 54.0.3, il 54.0.5 e il 54.0.6), nell'indifferenza generale, salvo una sacrosanta protesta da parte del presidente dell'8a Commissione, il senatore Grillo, che poco fa è intervenuto per farci una dottissima disamina sulla situazione di crisi economica, dimenticandosi però di ricordare quanto ha protestato all'interno della Commissione bilancio per quegli emendamenti, che, per sua stessa definizione, sono corposi emendamenti, che mettono mano in maniera incisiva alle norme che regolano un settore delicato quale quello dell'autotrasporto, cambiando regole, limiti ed obblighi. In meglio o in peggio

passino silenziosamente e surrettiziamente, approfittando del comodo autobus di una legge della quale, peraltro, si sa già che verrà blindata con un voto di fiducia. Qualcuno mi sa dire perché norme sui tempi per il carico e lo scarico delle merci debbano essere proposte all'interno di una manovra finanziaria? Qual è il beneficio che ne trarrà la finanza pubblica? Quali ricadute positive esse avranno sull'economia nazionale? Come diceva un nostro illustre collega, siccome a pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca quasi sempre, mi permetto di pensare che questi provvedimenti non abbiano seguito il loro *iter* naturale, passando al vaglio della Commissione competente, perché non si voleva sottoporli ad alcun esame: così come sono entrati in Commissione devono uscire da quest'Aula. È un piccolo esempio, se volete, ma è l'ennesima riprova della quale francamente non si sentiva il bisogno, della considerazione in cui vengono tenuti da questo Governo e da questa maggioranza le Camere, i loro rappresentanti e le loro funzioni. Signora Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, svolgerò pochissime considerazioni in una circostanza, come quella nella quale ci troviamo, in cui ognuno di noi si sforza prevalentemente di dare dare un senso al funzionamento di questa istituzione e anche - perché no - al nostro ruolo e alla nostra funzione. È noto che il Senato è impegnato da più di un mese nell'esame di una manovra, esame che si è concentrato fondamentalmente in Commissione bilancio e che ci vedrà, con un voto di fiducia annunciato,

La seconda annotazione è che la buona stella alla quale si era affidato il Presidente del Consiglio quando affermava che in fondo la crisi era più un fattore psicologico che un fatto reale in realtà si è rivelata una stella cattiva o inesistente: è stata è stata una scelta sbagliata, dalla quale è disceso direttamente il consumarsi inesorabile di quell'avanzo primario che era stato faticosamente reimpostato dalla prima manovra economica del Governo Prodi. Ricordo che in base a quella manovra l'anno prossimo, nel 2011, avremmo dovuto registrare il pareggio di bilancio: ahimè, siamo molto lontani da tale traguardo e ancor più lontani da quell'obiettivo di riduzione del debito che é, come sappiamo, il peso preponderante che sta sulle nostre ali. Insomma, siamo dinanzi a questa situazione: gli altri Paesi hanno potuto sviluppare politiche pubbliche anticicliche perché, potendo contare su una finanza pubblica più sana della nostra, hanno messo in moto risorse per sostenere la crescita in una situazione difficile e recessiva; noi a questi strumenti non abbiamo potuto ricorrere perché non avevamo risparmio nella finanza pubblica. Certo, il risparmio lo fanno le famiglie, ma ovviamente non potevamo utilizzare il risparmio delle famiglie per sviluppare una politica anticiclica. Anzi, le famiglie generalmente hanno sviluppato al contrario un'azione molto protettiva dei loro risparmi in questi mesi, in qualche modo determinando una situazione ancora più difficile. l'Europa, che un tempo era la causa di tutti i nostri mali, con questa manovra è diventata salvifica: meno male che c'è l'Europa che ci dice quanto dobbiamo tagliare e di quanto dobbiamo correggere. finalmente sviluppiamo in quel livello istituzionale un'azione, che voglio qui sottolineare, positiva da parte del Governo italiano, che appartiene a quella schiera di Governi dell'Unione che spinge per la realizzazione degli *eurobond,* e quindi perché si vada verso un bilancio dell'Unione europea che abbia la capacità di sviluppare azioni politiche indispensabili e necessarie in una fase come questa, senza ricorrere a interventi straordinari che si sono verificati nei confronti della Grecia, che ha visto tutti i Governi disponibili mettersi le mani in tasca per dare qualcosa per aiutare quel

Io appartengo a quella schiera di parlamentari e di politici che pensano che il federalismo non è mai stato una questione di risorse e nemmeno oggi è questione di risorse. Quindi, non mi iscrivo a quella schiera di coloro che affermano che con questa manovra abbiamo ammazzato il federalismo. Non è così! Il federalismo è una questione prima di tutto politico-istituzionale e la crisi del federalismo semmai va letta nei comportamenti che il Governo sviluppa quando nella

sul quale vorrei in futuro aprire una discussione più libera, con i nostri colleghi della Lega che si sono intestati il federalismo ma che stanno sostenendo decisioni del Governo che lasciano intravedere un futuro quanto meno più difficile per il federalismo

Abbiamo iniziato la nostra attività legislativa con il famoso decreto-legge n. 112 del 2008, che ha anticipato la finanziaria sul quale poi è stata puntualmente posta la fiducia. Abbiamo discusso la finanziaria, stiamo discutendo questa manovra, con i caratteri che ho ricordato. se siamo messi di fronte ad una proposta del Governo che si può o prendere o respingere, senza poterla minimamente valutare, avanzo una riflessione a tutti noi:

è una sua libera scelta, ha il conforto della maggioranza degli italiani. Ma l'opposizione non vi ha rinunciato: quindi, vorrebbe evitare di ritrovarsi nel corso delle prossime occasioni sempre davanti ad una manovra, «prendere o lasciare» senza che vi siano regole istituzionali che informino questa procedura, come per esempio avviene in altri Paesi. *(Applausi Signora Presidente, intervengo come parlamentare cialtrone di «Io Sud», in difesa di un Mezzogiorno tagliato fuori dalla manovra. Come parlamentare eletta capolista del PdL nel 2008, quando ci si presentò agli italiani con un programma, con un patto, cioè con un con la scheda n. 5, che ho sempre qui con me, nella quale si diceva: «Noi vogliamo un'Italia che finalmente superi attraverso un impegno straordinario il drammatico divario tra Nord e Sud, realizzando una politica che valorizzi la responsabilità dei territori e metta a frutto tutte le energie presenti nel Paese». E si declinava un piano decennale straordinario concordato con le Regioni per il potenziamento di porti, reti stradali ed autostradali, creazione di zone e porti franchi, addirittura leggi-obiettivo speciali, concentrate sul turismo, beni culturali, agroalimentare, risorse idriche, logistiche, infrastrutture, poli di eccellenza per la ricerca e l'innovazione, realizzazione di un piano strategico di riconversione dell'industria chimica pesante, pieno e tempestivo utilizzo dei fondi comunitari, realizzazione della Banca del Sud. Ma a questo dedicheremo poi un capitolo a parte, se e quando dovesse arrivare. Ebbene, questo patto avevo sottoscritto con gli italiani, con questa scheda n. 5 dell'obiettivo Mezzogiorno. Ho creduto all'epoca a quel patto, ma è stato tradito, non da me: è stato tradito da chi pensava di averlo sottoscritto con gli italiani. Quindi, se qualcuno si deve dimettere, come qualche collega meridionale del PdL dice, non sono certamente io, che non ho tradito il patto, ma sono gli altri che non lo hanno rispettato. È cominciata da subito l'espropriazione sistematica delle risorse per il Meridione, a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008,

Oggi con questa manovra, che si continua a ripetere essere in linea con la volontà dell'Europa, di fatto si attua solo la volontà del Governo di dividere l'Italia, contro la volontà vera dell'Europa che, se ricordo bene da ex parlamentare europeo, è quella di finanziare le politiche di coesione, di raggiungere l'obiettivo convergenza, di consentire cioè che le Regioni meno sviluppate si mettano al passo con quelle più avanzate.

sollevando il problema dell'aumento del divario tra regioni italiane. Partita questa manovra con la pretesa del rigore e dei sacrifici per tutti, alla fine ha rappresentato una sorta di cavallo di Troia per far passare con emendamenti blindati provvedimenti provvedimenti su cui il Parlamento avrebbe voluto semplicemente esprimersi. Penso al sistema pensionistico, piuttosto che alla riforma dell'autotrasporto. era partita con i grandi tagli che si sarebbero dovuti fare alla politica e si è immediatamente arresa alla richiesta - o meglio alla volontà determinata - della Lega di non tagliare neanche le Province: altro che Carta delle autonomie! Ci si è bendati gli occhi di fronte alla nostra richiesta non tanto di sopprimere un Ministero dell'agricoltura, teoricamente già soppresso per *referendum* per tre volte

una manovra che non esito a definire sprezzante anche solo nella forma. Penso all'articolo 4 intitolato impropriamente «Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni», che contiene invece la mini-naja e qualche milione di euro, non so se per le celebrazioni dell'unità d'Italia o per la secessione e la celebrazione della neonata Padania; all'articolo 15, nel quale, sotto la voce «Pedaggiamento della rete autostradale ANAS», si prorogano le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per ben sette anni e a condizioni assolutamente immutate. In tutto questo, ed altro ancora, il Mezzogiorno dov'è? Si prorogano pesantissimi sgravi alla città di Asti (ma non è assistenzialismo, naturalmente!) per l'alluvione del 1994. E poi non si ha voglia neanche di riconoscere lo stato di crisi per calamità atmosferiche a qualche regione che ha il semplice torto di trovarsi nel Mezzogiorno d'Italia. E addirittura, da parte di Governo e maggioranza, si soffre tanto per concedere agli abruzzesi la sospensione, o meglio lo slittamento dei versamenti tributari solo fino al 31 dicembre 2010. È una manovra che rappresenta una vera e propria beffa per i meridionali, a meno che qualcuno non pensi di far passare per interventi di favore per il Mezzogiorno l'aver inserito - nientemeno - l'acquisto del famigerato termovalorizzatore di Acerra, concedendo di poterlo acquistare con fondi regionali FAS. Poi qualcuno ci spiegherà che urgenza c'è di far acquistare alla Regione Campania il termovalorizzatore di un privato; o che senso ha aver scelto, tempo addietro, di concedere 500 milioni di euro per il dissesto di Catania senza avere pensato che forse un analogo provvedimento ci sarebbe potuto essere anche per il dissesto della città di Taranto. Ma la beffa continua con l'articolo 40, intitolato «Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno» dove, con un'ingerenza notevole dello Stato sulle autonomie, si concede, si fa per dire, alle Regioni del Sud di potere nientemeno che azzerare l'IRAP con una legge regionale, bontà del Governo. Ma non sappiamo che ci sono i commissariamenti per la sanità e che almeno quattro Regioni sono obbligate per legge dello Stato ad aumentare le tasse? E laddove dovessero azzerare l'IRAP, con quali entrate dovrebbero provvedere a tentare di garantire i servizi ai cittadini? Bene fanno le Regioni a protestare con decisione, ancor più le Regioni meridionali. Penso alla mia Puglia, che ha una sola certezza: un taglio di 287 milioni nel 2011, di 422 nel 2012 e addirittura di 597 nel 2013; e dovrebbe anche, bontà vostra, azzerare l'IRAP? Così vivremmo, come si dice dalle mie parti, di sole, di mare e di vento. intitolato «Rifinanziamento del fondo infrastrutture» mi aveva fatto sperare, perché pensavo si trattasse della famosa perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno. Invece no, tutto è subito messo in chiaro. Per i 635 milioni recuperati dai mutui della Cassa depositi e prestiti c'è una priorità chiaramente indicata con nome, cognome e indirizzo: 400 milioni di questo finanziamento sono per il MOSE, che notoriamente non è nel Mezzogiorno d'Italia ma nella laguna veneta, il resto chissà. Ma sì, tanto le imprese del Sud si dice che non funzionano, che non sanno andare avanti, che rubano, ed è noto, infatti, che il ponte sullo Stretto di Messina sarà realizzato da Impregilo, notoriamente con sede nel Mezzogiorno d'Italia. Così come meridionali sono certamente le imprese che da anni stanno tentando di costruire la Salerno-Reggio Calabria. Il Sud, quindi, non ha priorità. L'articolo 41 è poi titolato: «Regime fiscale di attrazione europea»: una bella cosa veramente, investimenti nel Mezzogiorno. A fronte di piccole e medie imprese, di aziende agricole meridionali, dunque italiane, che chiudono, perché non riescono a sopportare un pesante regime di imposizioni fiscali, un costo del lavoro eccessivamente alto rispetto agli scarni profitti, o che vengono addirittura vendute all'asta dalla usuraia Equitalia, si prevede di applicare alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea che, bontà loro, vogliono investire da noi, la normativa tributaria vigente in quegli Stati.

altro che attrazione di investimenti! Ma il massimo della beffa, o forse - diciamolo come va detto - del disprezzo nei riguardi del Mezzogiorno l'avete mostrato quando avete costretto il relatore (perché mi rifiuto di credere

fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno ed emendamento per le quote-latte. Avete poi bocciato per un voto, colleghi meridionali di maggioranza, una richiesta sacrosanta e legittima degli agricoltori meridionali, che chiedono soltanto conteggi corretti e veritieri da parte della previdenza sociale per poter procedere alla rateizzazione del loro debito dal Gruppo PD e del senatore D'Alia).* Ebbene, avete detto no a chi chiede di rientrare nella legalità. Avete detto un abbondante sì a chi continua ad evadere e a infischiarsene della legalità, dell'Europa, delle condizioni complessive dell'Italia. Ma certo: tutto regge, tutto ha una sua logica anche se, per me, è una logica perversa. Il figlio del ministro Bossi, nel suo comizio, aveva reso nota la promessa del papà sulle quote latte. *Pacta sunt servanda* l'ex ministro Zaia si è precipitato in Senato per garantire che l'emendamento potesse passare. Avrà avuto certamente qualche sua buona ragione. un collega della Lega, nel suo intervento, è stato onesto e chiaro nel ricordare che la Lega è nata con una missione precisa, alla quale non intende rinunciare. Ho annotato le sue parole: ribadito che tale missione era di raggiungere la libertà e l'indipendenza della Padania. Egli ha ricordato, per analogia con il Nord Italia, le vicende della Scozia, Scozia, ritenendo normale e legittimo l'insediamento di Ministeri a Milano, piuttosto che a Torino. Dunque, se le parole hanno un senso, questa manovra è dichiaratamente secessionista perché rappresenta un percorso chiaramente tracciato dal Governo,

ma tiene in un disegno politico che nulla ha a che vedere con la tanto proclamata e celebrata unità d'Italia. È proprio per tutto questo che è nata la componente «Io Sud»: non certo per agevolare la secessione, ma per riacquistare, da italiani, l'orgoglio meridionale. Porteremo noi in Europa questo comportamento assurdo e antiunitario dell'Italia e lasceremo a voi la responsabilità, nei riguardi degli italiani tutti, e degli italiani meridionali in particolare, di votare una manovra che, se avessi voluto usare un linguaggio pesante ma ormai in voga, avrei potuto definire cialtrona. Preferisco, però, definirla semplicemente secessionista e antiitaliana e chiedere ai colleghi tutti di esercitare nel voto quella libertà ancora teoricamente consentita agli eletti. Sentitevi eletti e non nominati: rappresentiamo l'Italia e, nell'Italia, i nostri territori e le ansie delle nostre genti. Riacquistiamo, con un voto libero e onesto, la nostra dignità di parlamentari. *Pacta sunt servanda* anche nei riguardi del Meridione.

darò qualche elemento di valutazione della manovra, almeno così come la conosciamo a questa mattina. Ciò rende un po' surreale questo dibattito, perché discutiamo di un testo che poi dovrà essere rimodificato nell'annunciato maxiemendamento. Questa però può essere un'opportunità, perché questo dibattito potrebbe, in qualche modo, trovare una misura d'ascolto da parte del Governo e del relatore, magari per inserire nel maxiemendamento elementi importanti di rafforzamento e correzione della manovra. Concluderò con l'illustrazione dello schema logico di un pacchetto molto piccolo, composto da 15 emendamenti che ho presentato a mia firma insieme ad altri 14 colleghi senatori, cercando di puntualizzare almeno tre o quattro aspetti di quello stesso pacchetto di emendamenti. Parto dalle due premesse. La prima riguarda riguarda l'entità della crisi e quella della manovra. Ricordo che nella scorsa sessione di bilancio, quindi sei mesi fa, avevo avuto modo di esprimere un'opinione, cioè la necessità di una manovra strutturale, riformatrice, che avevo quantificato in circa 35 miliardi di euro, addizionali rispetto alla manovra *soft* che era stata presentata in Parlamento. In quel momento questa proposta fu considerata cervellotica, mi fu attribuito il ruolo del dottor Stranamore, anche se non ho trovato negli elementi di confronto valutazioni che entrassero nel merito di quelle proposte. Vorrei far notare, signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, che da dicembre ad oggi quest'Aula e il Parlamento hanno dovuto occuparsi di tre manovre: la legge finanziaria, partita con un'entità di 5 miliardi e chiusa con un'entità di 9 miliardi; il decreto mille proroghe, all'interno del quale vi era il gettito *una tantum* dello scudo fiscale, che ha determinato una seconda manovra da 9 miliardi, e la manovra attualmente in discussione presentata il 31 maggio, pari, come sappiamo, a 25 miliardi di euro. l'aritmetica ci conduce a constatare che se a dicembre una proposta da 35 miliardi di euro fu giudicata cervellotica e da dottor Stranamore, a maggio siamo arrivati a 9, più 9, più 25, cioè ad una serie di tre manovre per una entità complessiva - se l'aritmetica non è un'opinione - di 43 miliardi di euro. Questa è la prima premessa. La seconda premessa, signora Presidente, fa riferimento a un mistero italiano, che si prolunga da oltre trent'anni, che ha attraversato la Prima e la Seconda Repubblica e che ha attraversato decine di Governi e innumerevoli Parlamenti. Qual è il mistero italiano? Per trent'anni tutti noi - almeno quelli di una certa età e che hanno partecipato alla vita economica, sociale e politica italiana - ogni anno, puntualmente, ci siamo trovati di fronte a Governi di varie colorazioni politiche che proponevano mega tagli della spesa. Se facessimo la sommatoria, attraverso i giornali dell'epoca, di quante decine e centinaia di migliaia di miliardi di vecchie lire prima, e decine di miliardi di euro dopo abbiamo tagliato di spesa pubblica, arriveremmo vicini al valore del PIL. del PIL. Per trent'anni abbiamo tagliato la spesa pubblica e nel frattempo la pressione fiscale è aumentata di dieci punti. Non dimentichiamocelo:

abbiamo aumentato le tasse e abbiamo il terzo debito pubblico del mondo: qui l'aritmetica non può più aiutarci, perché il bilancio è fatto di entrate, di spese e di saldi. Se si tagliano le spese e si aumentano le tasse come mai abbiamo un tale debito pubblico? Ecco il trucco, signor Presidente. Ripeto, è un trucco trentennale, rispetto al quale chiedo alla politica di confrontarsi per cambiare metodo. Il trucco consiste nel fatto che tutte le manovre di questi trent'anni - compresa quella che stiamo discutendo - sono riferite a tagli sulle spese tendenziali degli anni futuri,

l'aumento della spesa pubblica. Noi qui, oggi e nei giorni prossimi, non decideremo di tagliare la spesa pubblica, ma di aumentarla, perché ciò che conta nell'economia è la spesa pubblica del 2009 e del 2010; per il 2011 non conteranno i tagli sui tendenziali di tale anno, ma conterà, dopo i tagli effettuati, quale sarà la spesa pubblica effettiva del 2011. Questo è il cambiamento di metodo che chiedo alla politica e alla responsabilità della rappresentanza politica, per smetterla di prenderci in giro, dopo trent'anni; e ciò non è responsabilità dei singoli Governi in quanto tali, ma collettiva, prima e seconda Repubblica comprese. Nei Paesi civili del mondo, quando il presidente Obama, o il Presidente degli Stati Uniti di turno, fa il messaggio alla Nazione e annuncia il *budget*, non parla di tagli tendenziali, ma dice semplicemente - giusto o sbagliato che sia

aumentate, perché proposte strategiche di politica economica non vengono neanche considerate, ma altri tipi di inserimenti sì. ciò consegue la seguente valutazione; la manovra ci dice che si taglia il *deficit* pubblico di 25 miliardi, e siamo tutti d'accordo sulla necessità e l'urgenza, anche perché è un patto pregresso, fatto a novembre con l'Unione europea, che nulla ha a che vedere con la crisi greca, poiché era un impegno precedente. Questi 25 miliardi si tagliano attraverso 15 miliardi in meno di spesa e 10 miliardi in più di entrate.

è che stiamo decidendo di aumentare la spesa corrente di 26 miliardi rispetto ad oggi, di ridurre di 3 miliardi gli investimenti pubblici e di aumentare di 45 miliardi le entrate. Se fate i conti, vi ritrovate il taglio di 22 miliardi. Questo è quello che stiamo facendo e, in tale contesto, c'è una stima di 9 miliardi per la lotta all'evasione: sacrosanta lotta all'evasione. Attenzione, però: quei 9 miliardi, per ben 4 miliardi nel biennio, sono riferiti al provvedimento che riguarda la non deducibilità delle imposte per le imprese, se in presenza di un contenzioso tributario. francamente che quella norma sia un po' folle, anche perché non c'è commisurazione tra potenzialità della compensazione ed entità del

Sono totalmente d'accordo con la rimozione di quella misura; mi chiedo però come si coprano i miliardi di euro agganciati a quella specifica norma. Per concludere,

la procedura è la seguente: si parte dal quadro tendenziale macroeconomico, se ne deriva l'andamento tendenziale di finanza pubblica, si fa la manovra di correzione e qui finisce la procedura. Chiunque di buon senso - non occorre essere economisti - capisce che

il valore del prodotto interno lordo, e troverete che esso è identico al centesimo di euro sia nell'andamento tendenziale sia nell'andamento programmatico. Il che vuol dire che le manovre di decine di miliardi di euro sulla finanza pubblica non hanno nulla a che vedere con l'andamento della produzione, dell'occupazione, dell'economia reale: la controprova di quanto sto dicendo È evidente quindi che questa manovra, urgente e necessaria, produce effetti di freno sull'economia che il Governo ha stimato in mezzo punto di PIL, la Banca d'Italia in un punto di PIL, se si sommano gli effetti sui due anni, il mio Centro Studi Economia Reale ha stimato in un punto di PIL. Ma, al di là dei numeri, è evidente che l'effetto di freno sull'economia riduce la potenzialità di

ma va fatta nel federalismo fiscale. Francamente, qualcuno deve spiegare cosa c'entra la cedolare secca con il federalismo fiscale. Nulla! È ovvio che possiamo metterla nella normativa in esame, e poi, nel federalismo fiscale, dire che il gettito proveniente da quella IRPEF nazionale è di competenza dei Comuni. Se si deve fare, perché non farla adesso? Chiudo sulle Regioni. Gli enti locali hanno visto un taglio dei trasferimenti orizzontali di 8 miliardi e mezzo. 8 miliardi e mezzo. Una delle nostre proposte è quella di dire agli enti locali che, invece del taglio orizzontale dei trasferimenti, si può fare un patto tra Stato, Regioni, Province e Comuni, con il quale loro si impegnano a bloccare la spesa dilagante che hanno avuto nella voce degli acquisti di beni e servizi. Se tale spesa si bloccasse al valore di quest'anno, il risparmio sarebbe di 11 miliardi, molto di più degli 8 miliardi e mezzo. Sarebbe un'operazione verticale mirata su quella voce, che risanerebbe anche le aree grigie tra economia e politica diffuse sul territorio e non sarebbe un taglio orizzontale.

Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, i recenti provvedimenti della maggioranza e del Governo nei confronti delle persone disabili si configurano - dobbiamo dircelo - come un attacco vero e proprio ai loro diritti, sanciti dalla Costituzione, dal quadro legislativo nazionale ed europeo, nonché da importanti convenzioni dell'ONU. L'attacco ai diritti delle persone disabili non si ferma neanche quando queste persone sono bambini.

o comunque tutti si devono sacrificare, anche i disabili. Questo modo di ragionare, oltre che inaccettabile, è profondamente sbagliato e contrasta con il quadro legislativo. L'ultimo provvedimento è stato un emendamento presentato da due colleghi della maggioranza e accettato poi dalla Commissione; tale emendamento di fatto ha tolto il tetto dei venti alunni per le classi con bambini disabili.

«dopo aver rinunciato alle preannunciate disposizioni che avrebbero colpito le persone con disabilità (pensioni di invalidità, assegno di accompagnamento), ora» - con la Commissione bilancio del Senato - «rivolge la sua attenzione ai bambini, in una logica di apparente risparmio». C'è una contestazione puntuale di questa concezione del risparmio, perché è evidente che le classi sovraffollate richiamano gli insegnanti di sostegno e, siccome c'è il blocco, ci sarà il ricorso al giudice e quindi aumenterà moltissimo il contenzioso. Ma lo sdegno rispetto a questo emendamento passato in Commissione bilancio è stato espresso da moltissimi altri. Cito soltanto due persone, ma potrei citarne decine e centinaia: Giovanni Villarossa, dell'Unione cattolica italiana di insegnanti medi (UCIIM) e Nina Daita, della CGIL. Dice Giovanni Villarossa: «Suscita meraviglia, se non scandalo che qualche senatore abbia potuto pensare di risparmiare su un piccolissimo aspetto, che però procura grandissime difficoltà», perché in classi numerose diventa molto più difficile il processo di inclusione, anzi di integrazione scolastica degli alunni in difficoltà. che «è davvero una persecuzione, un'ossessione nei confronti del mondo della disabilità. Il modello di integrazione scolastica per le alunne e gli alunni con disabilità è unico in Europa ed apprezzato da tutti. Perché sgretolarlo? Vada per i sacrifici ma diciamo no alla discriminazione». che riconosce ai bambini italiani i propri diritti, specifiche forme di tutela e pari opportunità per lo sviluppo della loro personalità, autonomia e partecipazione sociale. Per quanto riguarda i bambini disabili, faccio riferimento alla legge-quadro

si è affermata anche nelle leggi di settore, passando dai bisogni di assistenza alle politiche di inserimento sociale, e a una considerazione non soltanto della disabilità, ma anche dei bambini disabili. le politiche innovative richieste riguardano le persone disabili in famiglia, il passaggio dalle strutture educative speciali a quelle ordinarie, la crescita e l'inserimento nella vita. In

l'assegnazione di un docente di sostegno per un tempo rapportato alla gravità della disabilità e la riduzione del

Fra le azioni migliori in una comunità che accetta di competere in Europa e nel mondo c'è anche quella che mette al centro della scelta le persone, il loro sistema di relazioni, l'opportunità per ciascuno di esprimersi al meglio. Ha commosso tutti quello che è successo in Spagna: i campioni hanno

signora Presidente. In queste ore i presentatori dell'emendamento hanno affermato che non intendevano

di adottare quelle scelte che consentano di raggiungere l'obiettivo di una migliore integrazione dei soggetti afflitti da disabilità. Questo è il risultato di un emendamento sbagliato, pasticciato, incompreso; c'è la possibilità di rettificarlo, come chiedono gli stessi presentatori, ed è è importante che ciò avvenga, perché i confini di civiltà non vanno toccati. Vorrei concludere con l'Italia che vorremmo, quella che non indebolisce i confini di civiltà costituiti dai diritti dei bambini disabili. Dice il poeta in una filastrocca per la Melevisione: «Tu non sei come me: tu sei diverso. Ma non sentirti perso. Anch'io sono diverso, siamo in due. Davvero ti son grato perché non siamo uguali: vuol dire che tutt'e due siamo speciali».

Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, è già stato ripetutamente ricordato negli interventi dei colleghi del Partito Democratico che mi hanno preceduto, a partire dalla relazione di minoranza del senatore Giaretta, che questa manovra correttiva non affronta nessuna delle priorità del sistema Paese ed, anzi, ne accentua le disuguaglianze aggravandone le condizioni, soprattutto in ordine all'erogazione dei servizi essenziali che in larga parte vengono predisposti, organizzati ed erogati su base territoriale. In questi pochi minuti vorrei parlare di ciò che accadrà in uno dei comparti, quello del trasporto pubblico locale, che ha ricadute consistenti su milioni di cittadini che da esso dipendono per l'organizzazione della propria vita quotidiana di lavoro, di studio, di impegno familiare. I tagli previsti per Regioni ed enti locali, che dovranno concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per 4,5 miliardi di euro, creeranno una situazione di scadimento e riduzione di questo servizio, a meno di non alzare le tariffe a livelli insopportabili soprattutto per le fasce della popolazione a reddito medio-basso: pendolari, lavoratori e studenti, in particolare. La manovra mette in discussione i 500 milioni di euro, su base annua, che hanno consentito nel 2009 il rinnovo in quasi tutte le Regioni dei contratti di servizio di Trenitalia nel trasporto regionale. Il taglio che si prevede, e che deriva dalla mancata trasformazione dei trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale in compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, rappresenta oltre il 20 per cento dei trasferimenti destinati per questa attività alle Regioni e rimette in discussione i contratti appena rinnovati ed i livelli di produzione dei servizi. Sono a rischio le acquisizioni di nuovo materiale rotabile perché il meccanismo con cui sono state attivate "in autofinanziamento" da Trenitalia si fonda sui flussi finanziari generati nel periodo di validità dei contratti stessi. Certo che una smentita così clamorosa alle vittoriose tappe del federalismo di stampo leghista non poteva essere più eclatante! È a rischio almeno il 25 per cento dei servizi e con esso anche lo sviluppo e la diffusione del trasporto pubblico locale in termini di investimenti ed estensione del servizio, con i contraccolpi che si avranno sul territorio sul versante sia economico che sociale. Sul versante dell'occupazione anche le aziende pubbliche del trasporto locale rientrano nei vincoli di *turnover* previsti dal decreto. Si tratta del divieto di effettuare, dal 2011 al 2013, assunzioni a tempo indeterminato eccedenti il 20 per cento dei rapporti cessati nell'anno precedente, limite che sale al 50 per cento nel 2014 e al 100 per cento nel 2015. In molte aziende tali vincoli si applicheranno indipendentemente dalle loro condizioni ed esigenze produttive. Ciò spianerà la strada alla terziarizzazione in appalto di molte attività e determinerà un ricorso massiccio al subaffidamento dei servizi di trasporto pubblico. Invece di intervenire sul taglio degli sprechi rappresentati da un numero abnorme di consigli di amministrazione, posizioni dirigenziali sovrastimate, consulenze e forniture in un sistema rappresentato da oltre 200 aziende alle quali si aggiungono, con la loro ulteriore dote di costi e diseconomie, 600 aziende cosiddette private ed altre 400 artigianali, familiari e cooperativistiche, si adottano interventi indifferenziati che produrranno una riduzione dei servizi e dell'occupazione soprattutto a scapito dei giovani entrati recentemente in questo settore con le tante forme di lavoro atipico e precario. Entro il 2012, come prevede la normativa vigente, tutto il servizio dovrà essere affidato attraverso procedure di gara. A seguito degli effetti prodotti dalla manovra correttiva avremo sicuramente tre certezze: aumenti, anche consistenti, delle tariffe; peggioramento del servizio; condizioni di lavoro peggiori e più precarie. aumenti delle tariffe e il peggioramento del servizio si riverseranno in maniera prevalente sull'intera utenza rappresentata dai pendolari e dalle fasce più deboli della popolazione. Molto elevati e prevedibili sono i rischi di un insostenibile impatto in termini ambientali, soprattutto nelle aree metropolitane o urbane del Paese, a seguito del depotenziamento del servizio e degli investimenti sulla mobilità collettiva: chi può ricorrerà al mezzo privato, con le conseguenze che tutti possiamo immaginare in un sistema viario già saturo e insufficiente. Venerdì scorso vi è stato lo sciopero generale - questa volta unitario - di tutto il comparto dei trasporti dei trasporti per richiamare l'attenzione del Governo su questi problemi. Non ce ne siamo accorti perché abbiamo già una buona legge che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero in questo settore con grande rispetto per i diritti degli utenti. Hanno scioperato civilmente, garantendo i servizi essenziali, quegli stessi servizi che voi vi preparate a tagliare e a peggiorare, senza che nessuno sia in grado di sanzionare un comportamento così irresponsabile, con buona pace del ministro Sacconi che vorrebbe ulteriormente ridurre il diritto di sciopero per i lavoratori di questo comparto. Con questa manovra si dà un ulteriore impulso al declino del Paese, di tutto il nostro Paese. Ho cercato di esemplificarlo riferendomi ad un settore in particolare, ma, com'è stato ripetutamente detto e dimostrato, ciò potrebbe valere anche per altri settori vitali del nostro Paese, perché purtroppo questa manovra è informe e non risolutiva. Essa è la dimostrazione che avete i voti per approvare «la qualunque», ma continuate a non avere un progetto per guidare il Paese sulla strada della rinascita, sia economica, ma anche - permettetemi di dirlo - morale.

Anzi, sin da subito è apparso carente sotto il profilo politico, contraddittorio sul piano della distribuzione dei sacrifici, incongruo ed inefficace rispetto ai risultati che dice di voler perseguire. Sotto il profilo politico si tratta del solito ricorso ai tagli lineari, cioè ad un meccanismo sostanzialmente automatico che impedisce di guardare dentro ai tagli che si effettuano e di premiare atteggiamenti virtuosi o penalizzare comportamenti scorretti; un meccanismo che vieta di compiere delle scelte, esattamente il cuore di ogni politica e di ogni azione di Governo fare delle scelte nell'allocazione delle risorse disponibili. Con i tagli lineari, effettuati in maniera cieca ed indiscriminata, si finisce per non scegliere, per non decidere, per non governare. Sul piano della distribuzione dei sacrifici - ed in tempo di presunta applicazione del federalismo fiscale - risulta incredibile il peso che la manovra consegna agli enti locali e alle Regioni rispetto a quanto riserva al Governo centrale: due terzi dei tagli gravano sugli enti locali, mentre all'interno delle Regioni - come al solito - si ritrova una sperequazione fortissima tra il Mezzogiorno Il peso economico di cui dovranno farsi carico le Regioni a statuto ordinario del Sud è di 211 euro *pro capite*, contro il Centro, che pagherà 194 euro *pro capite*, ed il Nord, che pagherà 129 euro *pro capite*.

Dei 10 miliardi che interessano le Regioni (8,5 miliardi le Regioni a statuto ordinario e 1,5 quelle a statuto speciale), solo per i trasporti la Calabria pagherà 283 milioni di euro;

Finiremo per arrivare a 1.250 milioni di euro: ben oltre un decimo dei tagli che saranno pagati dalle Regioni saranno a carico della sola Regione Calabria.

Venisse presto il federalismo fiscale se dobbiamo continuare con questo modo di governare un territorio che ancora - grazie a Dio! - è unitario. Probabilmente

manca del tutto l'intero pilastro indispensabile ad una seria manovra finanziaria; manca l'altra gamba senza la quale l'intera impalcatura non si può reggere. È quasi una legge fisica. Mancano tutte le misure necessarie per sostenere un minimo di domanda indispensabile per evitare che la manovra abbia solo l'effetto di deprimere lo sviluppo e la crescita del Paese. Ma non bisognava impressionare troppo gli italiani. Non bisognava evidenziare troppo che sono i finiti i tempi di Robin Hood e che, invece, la realtà è diversa e richiede sacrifici concreti e significativi. Se dovesse continuare la crisi si tratterà, probabilmente, di dover mettere mano ai modelli che riguardano il tenore di vita delle nostre società occidentali, troppo impegnate a vivere a debito, al di sopra delle loro possibilità e in un crescente imporsi di una logica tipica dell'esclusivo consumismo. Ed in questi scenari avremmo necessità di rafforzare le nostre garanzie nella consapevolezza che fenomeni come la globalizzazione - capace anche di essere l'*humus* dentro cui esplode la crisi non si possono solo demonizzare. Non si devono demonizzare, come, ad esempio, fa il Ministro del tesoro, perché dentro la globalizzazione, dentro i problemi e, se volete, insieme alla crisi che la globalizzazione ha amplificato, ci sta anche - guarda caso - la fuoriuscita dalle condizioni di povertà di qualche miliardo di esseri umani in qualche parte di questo nostro mondo. Proprio per questo, per non subire la globalizzazione, ma per starci dentro con determinazione e autonomia, dovremmo rafforzare le nostre garanzie. Dovremmo rafforzare il nostro Paese nella sua unità oltre che nella sua unicità, e dovremmo rafforzare la nostra Europa. Altro che diritto alla secessione, altro che quote latte o altro che quote latte o Ministeri sminuzzati di qua e di là! Questa manovra dimostra in maniera inequivocabile che non ci sono le risorse per realizzare il federalismo. Tremonti questo lo sa bene ma, consapevole che su questo finirà per implodere definitivamente l'attuale maggioranza, deve tenerlo nascosto agli elettori della Lega Nord e minimizzare. Purtroppo si tratta di questo, ed è per tale motivo che sono stati scartati e respinti tutti i suggerimenti emendativi migliorativi di quanti, pur dall'opposizione, si preoccupano delle sorti del nostro Paese. Noi abbiamo provato a dare una mano, lo abbiamo fatto attraverso 26 emendamenti alla manovra pensati per affrontare i nodi strutturali e recuperare oltre 5 miliardi di euro. Intanto, partendo dai costi della politica. È strano come tutti i soggetti siano chiamati a partecipare alla crisi, a fare sacrifici, tranne i partiti politici percettori di finanziamenti pubblici. Avevamo chiesto, come ApI, di ridurre del 50 per cento il finanziamento alla politica fin da subito e sopratutto di mettere fine a quello scandalo secondo il quale la politica si finanzia anche autoattribuendosi voti non espressi dagli elettori. Spesso volutamente non espressi. Avevamo chiesto di mettere mano seriamente al taglio di quelle Province oggettivamente inutili, ma non abbiamo avuto ascolto. Così come non abbiamo avuto ascolto quando, con precise proposte emendative, ci siamo chiesti se era possibile richiedere un sacrificio, così come facciamo per esempio per gli insegnanti dei nostri figli, anche a quei nostri connazionali che hanno "scudato" parte dei loro beni: una quota straordinaria, un 5 per cento a titolo di imposta straordinaria e di solidarietà, destinando il 50 per cento del ricavato alla diminuzione del debito pubblico e l'altro 50 per cento a finanziare il settore della formazione (scuola, università, cultura e ricerca). Niente da fare. Avevamo chiesto che gli intermediari intervenuti nella fase di regolarizzazione in base allo scudo fiscale garantissero circa la congruità dei beni coperti dallo scudo, in particolare per le società con sede all'estero che possiedono patrimonio immobiliare in Italia. Così come anche noi avevamo chiesto fin da subito l'introduzione della cedolare secca sugli affitti o lo scorporo e la liberalizzazione della rete del gas. Per non parlare delle questioni che riguardano la *green economy,* dai certificati verdi al trasporto locale.

Due emendamenti, poi, riguardavano proprio il federalismo fiscale: uno prevedeva la sospensione dell'attuazione dei decreti delegati della riforma quando la crescita annuale del PIL è inferiore all'1 per cento; l'altro prevedeva una sospensione fino a quando non saranno definite le misure di copertura del decreto attuativo sui tributi locali. Solo su un punto abbiamo avuto ascolto, ed esprimiamo la nostra soddisfazione ed il nostro ringraziamento anche al Presidente della Commissione bilancio. Un nostro emendamento è stato approvato: si tratta di una proposta che mette una stretta alle false dichiarazioni di invalidità dopo un incidente stradale per riscuotere i risarcimenti delle assicurazioni. Quello dei falsi invalidi è un cavallo di battaglia mulinato per screditare il Sud. Gli altri fanno chiacchiere, noi facciamo fatti. Alleanza per l'Italia è riuscita a proporre questo emendamento e a farlo approvare in Commissione bilancio punendo quei medici che attestano falsamente uno stato di micro-invalidità conseguente ad un incidente stradale per ottenere il risarcimento da parte delle società assicurative. È un provvedimento che mira ad eliminare un fenomeno di illegalità, che costringerà le assicurazioni ad abbassare le tariffe. Tuttavia, nonostante la nostra soddisfazione per questo emendamento,

*(PD)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, fin dall'inizio della legislatura il Gruppo del Partito Democratico, attraverso un'azione seria e responsabile, in Commissione agricoltura come in Aula, ha sollevato il problema della sofferenza del comparto agricolo, chiedendo consistenti misure di sostegno ed interventi adeguati a favorirne il rilancio e la competitività, naturalmente della sua rilevanza sotto il profilo economico ed occupazionale, nonché allo scopo di promuovere meglio le sue eccellenze nel mondo. Non vi è stato provvedimento, tra quelli utili a tal fine, che non abbia trovato il puntuale richiamo del Gruppo del attraverso la presentazione di emendamenti e la insistente richiesta al Governo e alla maggioranza di non disattendere le istanze del comparto. Abbiamo registrato, a fronte di grandi proclami, che soprattutto durante la presenza del ministro Zaia al Governo hanno trovato il loro momento di massima espressione nella comunicazione mediatica, soltanto promesse mancate. Rendo con qualche esempio quanto ho appena affermato: stabilizzazione delle agevolazioni contributive delle zone svantaggiate e montane; finanziamento del fondo bieticolo-saccarifero; agevolazioni relative all'uso del gasolio per le coltivazioni in serra; fondo investimenti in agricoltura; Fondo confidi regionali; credito d'imposta per l'internazionalizzazione in agricoltura; sostegno all'impresa giovanile e femminile; Fondo di solidarietà per i danni alle colture provocati da calamità naturali. Ci saremmo attesi che almeno in questa circostanza, e cioè quando si è finalmente preso atto dell'esistenza della crisi economico-finanziaria anche in Italia, si disponessero provvedimenti convincenti e rispettosi delle esigenze del comparto e della dignità professionale di quanti vi operano. Ed invece la manovra anticrisi del Governo penalizza fortemente l'agricoltura, le politiche agroalimentari e della pesca: alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», la riduzione relativa alla missione relativa alla missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" è di 3.880.000 euro per il 2011 e di 3.746.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Inoltre, la voce del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali evidenzia tagli complessivi di oltre 23 milioni di euro per il 2011, circa 18 milioni per il 2012 e altrettanti per il 2013. Su una riduzione totale di 58,2 milioni di euro in tre anni, oltre due terzi riguardano investimenti. Bisogna poi sommare i tagli già operati in sede di approvazione del bilancio e della finanziaria 2010, che avevano già prodotto la riduzione di un quinto degli stanziamenti (cioè meno 20 per cento) rispetto al 2009.

Emblematico a tal proposito è il caso della stazione sperimentale di Parma per l'industria delle conserve alimentari (SSICA) di cui è prevista la soppressione. Lo Stato non spende un centesimo per sostenerla, in quanto i contributi pubblici sono azzerati già dal 2009 e dunque la stazione sperimentale in questione si regge con il concorso dei privati, in particolare delle imprese conserviere, che versano contributi obbligatori attraverso le rispettive cartelle esattoriali. Ma c'è di più. Ad Angri, in

attraverso la previsione del decreto-legge n. 78, il centro di Angri dipenderà dalla camera di commercio di Parma. È incredibile, ma è così! Lo stesso comma 20 dell'articolo 7 prevede parimenti la soppressione dell'INCA (Istituto nazionale conserve alimentari), senza badare che con legge n. 99 del 2009 l'INCA era già stato soppresso e con decreto di riordino del 23 aprile 2010 è stata sancita l'eliminazione delle sue funzioni residue. L'INCA viene dunque "resuscitato" e subito soppresso aggregandolo all'INRAN e vanificando il lavoro di oltre un anno teso ad alleggerire il settore conserviero dal punto di vista economico-finanziario

evidentemente utile a ripianare almeno in parte il deficit dell'INRAN. Noi crediamo che tale soluzione non sia altrettanto utile a garantire la prosecuzione dell'attività in un settore molto delicato come quello della certificazione delle sementi, cioè dello strumento peculiare per garantire l'agricoltura di qualità. Tutto ciò in totale spregio del parere formulato dalla Commissione agricoltura del Senato, che ha espresso unanime contrarietà in ordine alla soppressione dell'ENSE e delle stazioni sperimentali per l'industria, con particolare riguardo a quella per le conserve alimentari. La chiusura del Governo e del relatore è incomprensibile ed è sintomatica di un atteggiamento di preconcetta ostruzione anche alle richieste - come questa - più facilmente come questa - più facilmente accoglibili, in quanto prive di effetti sulla spesa. Io sono francamente indignato per la sordità e l'insensibilità manifestata, oltretutto introducendo nell'emendamento 7.2000 del relatore in proposito due pesi e due misure; solo l'ENSE è fuori, mentre per gli altri enti soppressi è previsto un rinvio al decreto legislativo che stabilirà

ai Resoconti della seduta - la percezione netta di una noncuranza della sofferenza del settore primario da parte del Governo, purtroppo assecondata dalla maggioranza - e lo dico con estremo rammarico per mera necessità politica. E questo accade mentre si registra una situazione veramente preoccupante, se è vero come è vero che il calo dei redditi agricoli in Italia nel 2009 è risultato del 25 per cento, cioè esattamente il doppio rispetto al 12,5 per cento dell'Unione europea. L'Italia è il secondo Paese ad aver subito un così massiccio calo del reddito agrario. È preceduto solo dall'Ungheria! La riduzione dei margini e degli incassi ha determinato difficoltà nei pagamenti alle banche: l'agricoltura, come evidenziato dall'ABI in una recente audizione al Parlamento, rischia di tornare nella lista dei settori ad alto rischio dì solvibilità, in quanto fa registrare una crescita delle sofferenze bancarie.

Il mio intervento affronterà il rapporto tra la manovra e il federalismo fiscale, argomento piuttosto dibattuto, con opinioni in materia anche piuttosto diverse. Penso che sia innegabile il contrasto, netto e molto profondo, tra la direzione nella quale va questa manovra e la legge che abbiamo approvato lo scorso anno in materia di federalismo fiscale, che attua l'articolo 119 della Costituzione. Innanzi tutto, c'è un problema di rapporto tra le varie componenti della Repubblica, e quindi il Governo centrale, le Regioni, le autonomie locali. A parte l'accordo che è stato fatto tra Governo e Comuni, ma che comunque non rappresenta un avallo dei Comuni alla manovra, sulla quale mantengono un forte giudizio critico,

anche per proporre quelle riduzioni di spesa che sono necessarie nel momento in cui dobbiamo contribuire tutti quanti ad una minore spesa pubblica perché ci è chiesto dalla contingenza finanziaria ed economica internazionale. C'è però un problema molto serio per quanto riguarda i pesi. Anche qui ci sono dei dati inequivocabili, pubblicati nel recente rapporto sulla finanza pubblica italiana che precisano che il peso di tutta la spesa locale (quindi, compresa anche quella delle Regioni) sul complesso della spesa pubblica, al netto degli interessi sul debito, è del 31,6 la manovra pesa per il 2011-2012 per ben il 60 per cento sul comparto Regioni ed enti locali, percentuale che agevolmente aumenta fino al 65-70 per cento se consideriamo anche gli effetti dei tagli lineari sulla spesa dei Ministeri centrali che si ripercuotono poi su risorse trasferite ad enti locali e Regioni. Quindi, siamo di fronte ad un ribaltamento netto. Per essere equa dal punto di vista istituzionale, la manovra avrebbe dovuto essere costruita a rovescio; quindi, si tratta sicuramente di un eccesso di peso della manovra sugli enti locali che non si spiega.

nel 2011, 2012 e 2013 si apporteranno dei tagli che saranno poi neutrali ai fini dell'applicazione della legge sul federalismo fiscale. Cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui quella legge diventerà operante si presuppone che questi tagli vengano restituiti. È ovvio che ciò non è possibile perché siamo in condizioni tali per cui ciò non potrà accadere. Qual è allora il ragionamento che sta sotto a tutto ciò?

comporterà una riduzione di spesa, perché è evidente che tutti saranno tenuti a rendere servizi alla media più efficiente, tali riduzioni di spesa saranno assorbite dal Ministero dell'economia e saranno sostanzialmente il saldo della manovra che adesso viene proposta. tutto questo vuol dire minori risorse al sistema delle Regioni e delle autonomie locali, ma soprattutto vuol non rispettare la legge n. 42 del 2009. Noi del Partito Democratico abbiamo contribuito a quella legge, coerente con lo spirito della Costituzione, soprattutto perché prevede un federalismo solidale e cooperativo che va ad aumentare, con il patto di convergenza, l'offerta di servizi sui territori che ne sono meno dotati. Faccio presente anche - soprattutto ai colleghi della Lega, a cui il federalismo fiscale sta giustamente a cuore (e sta a cuore anche a noi) che parlare di autonomia impositiva come una sorta di araba fenice alla quale si potrà approdare dopo qualche anno di sacrificio, è parlare di nulla se quell'autonomia impositiva locale e regionale non viene finanziata, perché le varie leggi di stabilità stabiliranno anche qual è il livello della pressione fiscale complessiva. Quindi, o c'è la possibilità di finanziare quell'autonomia anche con la riduzione della spesa inefficiente oppure, ancora una volta, quell'autonomia non ci sarà, come oggi, perché ricordo che le aliquote, sia dell'addizionale IRPEF che degli altri tributi locali, sono bloccate. Ciò vuol dire che esiste una contraddizione profonda e insanabile, sulla quale noi, come Partito Democratico, ci riserviamo di essere molto precisi e molto netti nel nostro giudizio e, soprattutto in fase di discussione sui decreti legislativi delegati

che con queste norme stiamo violando la competenza e l'autonomia delle Regioni. Non si è mai visto che un Governo revochi gli atti adottati da una Giunta o da un Consiglio regionale: potrebbe infatti imporre altre misure nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica. Non si è mai visto che si revochino i contratti senza alcun indennizzo, perché ciò non è previsto dall'ordinamento vigente in Italia. Non si è mai visto che si disponga che i Comuni non possano costituire società miste all'interno di un certo parametro. assolutamente, che si possa procedere in questo modo dal punto di vista dell'efficienza e dei presupposti della necessità e urgenza, visto che poi si autorizza una giunta regionale (in questo caso quella della Campania) a fare otto assunzioni di *staff* per sfuggire

Il PD non lo ha mai discusso, perché è convinto che questa manovra fosse necessaria e ineludibile visto quanto accade dal punto di vista dell'economia globale, della crisi finanziaria, finanziaria, del rapporto tra debito e PIL (che in questi anni è fortemente cresciuto), per tutto ciò che ci obbliga a guardare oggi e anche in futuro sempre più alla necessità di considerare una disciplina dei vincoli di bilancio a livello europeo e mondiale, a rafforzare le regole delle cooperazione economica, ad aumentare la capacità di innovazione produttiva, a fare i conti con i consumi, con le materie prime, con il tema dell'energia, con l'evasione fiscale. E con il contrasto ai paradisi fiscali, con la bassa crescita che in questi anni in Italia si è determinata, con l'aumento nell'ultimo biennio del debito rispetto al PIL e dell'evasione fiscale. A tutto ciò aggiungiamo i dati strutturali di debolezza del nostro sistema Paese, compresa una mancata strategia sul Mezzogiorno, che non è solo un tema di risorse ma di riforme, anche se, ancora una volta, le risorse sono state sottratte. Ora, è evidente che la manovra era necessaria (l'hanno infatti varata tutti i Paesi europei), ma questa manovra avrebbe richiesto l'esercizio non solo del comando, ma del governo della complessità economica e sociale dell'Italia. E non si poteva eludere un confronto vero con l'opposizione, confronto che non c'è stato, quasi totalmente eluso, nonostante proposte di merito efficaci e alternative. La nostra contrarietà alla manovra nasce dal suo profilo, dalle scelte di fondo che sono stato fatte e da quelle che non sono state fatte. Questo provvedimento è stato definito iniquo; a mio avviso è insufficiente e, per qualche aspetto, perfino irrealistico dal punto di vista delle previsioni delle entrate. È vero che era necessaria una correzione dei conti pubblici e una riduzione del debito: ma questo basta? O era necessaria, in queste contingenze internazionali, una manovra che avesse il respiro non solo di una politica di bilancio, ma anche di una visione della politica economica di questo Paese? Era utile produrre tagli orizzontali alla cieca nel settore pubblico, indistintamente, senza individuare i fattori di rischio e di improduttività, che pure sono presenti? Era assolutamente necessario, forse, affrontare il tema della riforma della pubblica amministrazione, ma che fine ha fatto? Si è dissolta in un po' di "faccine", come ha detto il ministro Brunetta, o in qualche strombazzante annuncio. Magari si fosse davvero affrontato questo tema! Era Era necessario imporre vincoli centralistici, come alcuni colleghi hanno ricordato, che non hanno premiato il merito, la virtuosità di settori, di comparti, di Comuni, ma hanno depresso anche la capacità di mettere in campo risorse che potevano determinare la produttività e il lavoro sui territori? Era opportuno far pesare i sacrifici su fasce di popolazione già provate dalla crisi? Perché di fronte a questi fattori di rischio e a questi sacrifici non si è prospettata invece un'idea di futuro? Non si è affrontato il tema drammatico delle giovani generazioni. Queste generazioni, già attive dal punto di vista lavorativo, trovano difficoltà a costruire il proprio futuro; a queste generazioni si sta rubando il futuro, si stanno creando situazioni distorte dal punto di vista demografico, sociale, culturale. al permanere oltre un'età ragionevole nel nucleo familiare, all'impossibilità di crearsi una famiglia, oltre alle conseguenze psicologiche di chi vuole e deve guardare al futuro con fiducia, ha voglia di crescere e di progredire. Stiamo mortificando talenti, intelligenze, i beni e le merci più preziose che questo Paese ha: il capitale umano. Come risponde a tali interrogativi un Governo di centrodestra che negli ultimi nove anni ha governato Come ha affrontato tale tema in questa manovra, cosa che, invece, hanno fatto altri Paesi europei, compiendo, sì, scelte di rigore, ma anche di prospettiva? A queste domande non abbiamo trovato risposte; non abbiamo trovato soluzioni, da contrastare o da criticare, per la crescita e per lo sviluppo. Non abbiamo trovato quasi niente che dia il senso e il significato ad una manovra che appare di scarsa ambizione, che fa pagare prezzi sociali ed economici e che può creare, soprattutto in alcuni territori, fasce di esasperazione, oltre che individuali, anche collettive. Qualche segnale già appare e dovrebbe destare preoccupazione sociale. Ma chiedo a voi tutti, che pare vi apprestiate a votare questa fiducia, almeno annunciata per il momento: come si può chiedere ad un padre, ad una madre di famiglia, in questo quadro di difficoltà, di stringere ancora la cinghia fino all'esasperazione, talvolta fino alla perdita del posto di lavoro, se non si dà una prospettiva, se non si dà la possibilità di vedere almeno un lavoro per i propri figli, uno spiraglio di futuro? La crisi è sicuramente drammatica, ma nella crisi si misura la capacità di trovare prospettive; nella crisi si tiene insieme una comunità e un Paese; nella crisi bisogna evitare le lacerazioni, le divisioni, le chiusure e le difese corporative. È nella crisi che si esprime una guida che sia capace di far ritrovare tutti uniti in uno sforzo collettivo. Ma purtroppo di assenza di valori, di idee, di futuro e di prospettive questo Paese sta quasi soffocando e voi avete la responsabilità consistente che vi è stata affidata dai numeri, ma non dimostrate, credo, di essere all'altezza di questa sfida. Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, alcuni colleghi, soprattutto i senatori Mascitelli e Giaretta nelle loro relazioni di minoranza, hanno già espresso un punto di vista critico d'insieme su questa manovra. Fisserò l'attenzione soltanto su due punti. Il primo punto riguarda drammatica di finanziamento che viene riservata alla scuola, all'università e alla ricerca. Non sto a citare i numeri, perché ormai sono notissimi; si tratta di cifre impressionanti e crescenti nel corso degli anni, che impoveriscono il settore fondamentale su cui il Paese potrebbe cominciare a ricostruire una prospettiva di sviluppo. La scuola è impoverita, gli insegnanti diminuiscono, anche se non si capisce perché insegnanti di religione. Nell'università prolifera l'abitudine dei contratti a titolo gratuito; si chiede a ricercatori più o meno giovani, ma quasi tutti preparati, capaci e sperimentati, di occupare una parte sostanziale della loro vita, trasmettendo ciò che sanno, la conoscenza e la disciplina scientifica, gratis. Si immagina una riproduzione della conoscenza ed una trasmissione della capacità di ricerca sostanzialmente sulla base del lato volontario. Se ci state, lo fate, se non ci state, non lo fate; se nessuno lo fa, chi se ne frega. ciò fa pensare ad una sorta di rinuncia da parte del Governo a nutrire un settore fondamentale della società. Forse si pensa ad una privatizzazione, ma non si dice nemmeno questo. Sappiamo che il ministro Tremonti, che è così avaro di finanziamenti alla scuola pubblica, all'università ed alla ricerca, dedica i pochi soldi che ha ad una specie di istituto fantasma, che è l'Istituto italiano di tecnologia (IIT), di cui ancora si ignorano le prove ed i successi, ma che comunque è capace di ingabbiare parecchi soldi. Non sappiamo che fine essi faranno, ma sappiamo che questo IIT, che è una specie di scimmiottatura italica del Massachusetts Instituteof Technology

Il panorama è desolante. Non aggiungo altro; mi chiedo però come faccia il Governo a non rendersi conto che, se la trasmissione della conoscenza è affidata all'atto volontario di chi lavora gratis, gratis, forse noi siamo sull'orlo del baratro. Il secondo punto del mio intervento è molto particolare e speciale, ed è stato sollecitato da un'invenzione della Commissione, che all'articolo 49 ha introdotto degli emendamenti che, se letti alla lettera, sono veramente pericolosi: si tratta della trasformazione della dichiarazione di inizio attività in questa sorta di certificazione autodiretta dell'inizio attività.

e, in pratica, tutta la prassi che vuole il rispetto programmato delle disposizioni di piano paesistico e strutturale, del regolamento edilizio tutto il quadro - che per la verità, lo sappiamo, è barocco - dei meccanismi che presiedono al controllo del territorio viene sostanzialmente fatta fuori da una sorta di «liberi tutti» per l'impresa.

e si determina una situazione per cui l'ente pubblico, qualsiasi esso sia, ha solo 30 giorni per dirle di non proseguire poiché sta facendo un danno. Questa situazione ha qualcosa di inverosimile. Sappiamo che c'è un retropensiero costituzionale, dilettantesco e alquanto sgangherato, che immagina una revisione della Costituzione sulla base del fatto che l'impresa deve contare di più; mi riferisco alla revisione dell'articolo 41 e all'idea di santificare l'impresa, di cui francamente non si avverte il bisogno da alcun punto di vista. Nell'articolo 41 l'impresa è celebrata per quanto deve essere e la libertà d'impresa non è negata a nessuno. Si vuole stabilire il principio che l'impresa ad un certo punto può fare e, in nome del fare, far male. Viene svuotato il principio contenuto all'interno del codice dei beni e delle attività culturali, che porta perfino il nome del ministro Urbani. sulla base di questa prassi, perfino ciò che il centrodestra ha immaginato come gestione del territorio e del paesaggio viene annichilito per dare all'impresa la possibilità sovraordinata di di decidere la propria sorte a danno della sorte collettiva. In realtà, quell'emendamento

non sto a citare ma che sono di varia natura, si fermi sulla soglia, rinunci a portare questo colpo definitivo allo strazio del paesaggio italiano

Se pensiamo all'avidità dei «roditori privati» che si scateneranno sulla base di quest'emendamento, dobbiamo avere la lucidità di immaginare che gli enti pubblici dovranno rincorrere

Questa prospettiva ha qualcosa di angoscioso. Questa sarebbe la semplificazione? Questo sarebbe il criterio con cui diminuiamo il peso della burocrazia? Delle due l'una:

Dare addirittura il titolo di impero alle cose turpi che abbiamo visto accadere negli ultimi anni è veramente un elogio eccessivo della realtà. Queste compagnie

Usiamo le parole giuste. Gli imperi sono sempre qualcosa di più serio: leggete i classici. L'impero, se c'è, può essere oppressivo, può essere l'espressione di un potere assoluto, ma è qualcosa di diverso, e ha per lo meno qualche crisma di nobiltà. Qui la nobiltà che siamo costretti a vedere è la miserabilità dei sotterfugi e degli incontri al più basso livello degli affaristi peggiori, che corrompono la politica e la giustizia. I magistrati si vendono, i presidenti di Cassazione dicono: ora vado in pensione, e poi cosa faccio?

finestra"). È presente in tribuna una rappresentanza della Camera dei deputati della Provincia di Santa Fe, in Argentina, guidata dal presidente Edoardo Di Pollina. A loro va il saluto dell'Aula.

Illustre Presidente, egregi membri del Governo, onorevoli colleghi, prendo la parola quale rappresentante eletto - con oltre 20.000 preferenze nominali - nella ripartizione Europa della Circoscrizione estero per conto della lista «Berlusconi Presidente», nonché come delegato al congresso fondativo del Popolo della Libertà e come iscritto al partito, per confermare il sostegno parlamentare alla manovra in esame. La crisi nasce dalla finanziarizzazione dell'economia reale, fenomeno da noi denunciato in tempi non sospetti, ovvero già agli inizi di questo decennio, dalle colonne del «Pensiero londinese», il giornale della nuova emigrazione professionale di stanza a Londra. Le dinamiche globalizzate sulle quali le grandi banche d'affari della *city* facevano leva per attività di *trading* e di *merchant banking* evolvevano già allora con una velocità e complessità tecnica assolutamente superiori rispetto alle cornici regolamentari entro le quali avrebbero dovuto essere limitate. La politica occidentale ignorava, più o meno consapevolmente, il pericolo e devolveva all'autoregolamentazione, con l'auspicio che la «mano invisibile» del mercato supplisse in modo più efficiente alla mancanza di controlli efficaci. Fiumi di denaro finanziario scardinavano i precedenti argini normativi e illudevano legioni di amministratori, sia pubblici che privati, ignari delle conseguenze sociali delle loro adesioni alle proposte perfettamente presentate da alcuni banchieri. Il risultato sull'economia reale è stato devastante, specie in termini occupazionali. Fondamentali sono stati gli strumenti, quali la CIG ordinaria e straordinaria, utilizzati dal Governo per garantire la tenuta sociale del sistema Italia. Anche questa manovra va nella direzione di una opportuna revisione della spesa e di un raccordo più coerente con la situazione debitoria del nostro Paese sui mercati internazionali e, dunque, va sostenuta con convinzione, per scongiurare punizioni ancora più inique da parte degli speculatori internazionali. Sarà però compito non più procrastinabile del legislatore (sulla scia di quanto stanno facendo i colleghi parlamentari statunitensi e tedeschi, i primi a reagire concretamente) rimettere presto mano alla regolamentazione del settore finanziario, al fine di ricondurlo alla sua propria funzione di supporto all'economia e agli scambi, per non trovarsi di nuovo a breve nella paradossale ed immorale situazione - registrata in particolare nel Regno Unito di dover salvare i colpevoli con soldi pubblici, per ritrovarli intenti negli stessi perversi (ma per loro lucrativi) esercizi solo qualche mese dopo. Come emigrato all'estero (dal 1992) e come più giovane senatore della maggioranza, non posso peraltro non cogliere questa rara occasione per segnalare una forte anomalia del sistema Italia, che purtroppo anche questa manovra non sembra tenere in debita considerazione e/o correggere. Mi riferisco naturalmente alla cosiddetta emergenza occupazionale giovani e al fenomeno direttamente collegato della fuga dei talenti (secondo una felice espressione di Sergio Nava). In Italia è in atto un peggioramento consistente della condizione della fascia giovanile della popolazione, cioè delle persone con età compresa tra 18 e 29 anni. Il tasso di occupazione giovanile è sceso al 44 per cento, con una caduta tre volte superiore a quella subita dal tasso di occupazione totale. Una flessione, quella dell'occupazione giovanile, particolarmente brusca e repentina. E non c'è preparazione che tenga: nessun titolo di studio è stato in grado di proteggere i giovani dall'impatto della crisi. In particolare, i figli che vivono nella famiglia di origine, spesso impegnati in lavori temporanei e con bassi profili professionali all'inizio della loro carriera lavorativa, sono arrivati a rappresentare il gruppo più colpito dal calo dell'occupazione (meno 332.000 unità, secondo i dati ISTAT 2010). Nel 2003 la permanenza a casa era frutto di una libera scelta; adesso la prolungata convivenza dei figli con i genitori dipende soprattutto dai problemi economici. Per definirli è *not in education, employment or training* (non lavorano, non studiano, non si formano). I *neet* nel 2009 sono arrivati a oltre due milioni, il 21,2 per cento del *range* Il fenomeno mi tocca direttamente, oltre che per la giovane età, soprattutto per il fatto che molti giovani sono costretti dalla situazione sopra menzionata ad emigrare: oltre 40.000 l'anno, una vera e propria fuga di talenti. Quello che si vuole qui mettere in evidenza, però, è che le attuali generazioni di giovani italiani si trovano, senza colpe e loro malgrado, a dover scontare gli effetti concomitanti di diverse patologie della moderna società italiana. Tra queste vi sono, per sommi capi: il debito pubblico, la gerontocrazia, il sistema previdenziale e pensionistico, la mancanza di meritocrazia ed il dualismo del mercato del lavoro. Il debito pubblico, in particolare, accumulato dalle generazioni immediatamente precedenti, ha toccato il record di 1.827 miliardi e graverà sempre di più sulle nuove generazioni, penalizzando in modo inaccettabile i giovani italiani: è la prima volta che accade nella storia del nostro Paese. Viene minata la correttezza del rapporto intergenerazionale ed il principio giuridico e morale secondo il quale è tenuto a pagare il debito il soggetto che lo ha contratto. Per mancanza di tempo, deposito agli atti il documento più elaborato nel quale vengono identificate alcune proposte legislative ed esecutive concrete per affrontare l'emergenza giovani sopramenzionata. PRESIDENTE. La Presidenza ribadendo che nel nostro Paese è da tempo in atto uno scollamento generazionale a totale sfavore dei giovani e ciò avviene in vari campi (sociale, occupazionale, previdenziale e culturale); è la prima volta che accade nella storia della nostra Repubblica e non è giusto, né previdente; verifica per un *deficit* di rappresentanza (che è anch'esso parte del problema) facilmente verificabile, ma non per questo accettabile. Questi giovani, improvvidamente definiti bamboccioni, non hanno le possibilità che avevano i loro genitori, anzi devono pagare i loro debiti, sogneranno solo le loro pensioni e per lo più non riescono nemmeno a lavorare e mettere su famiglia perché il sistema è contro di loro. Addirittura, fanno concorsi durissimi e dopo non vengono assunti, come nel caso dei 107 dichiarati vincitori di concorso all'Istituto nazionale per tra 15.000 candidati, che non vengono assunti, o come altri nella stessa situazione all'INPS. Quali prospettive si prevedono per questi giovani? Molti, troppi, sono costretti ad emigrare e per loro e per loro la strada del ritorno è stata finora impossibile. È vero che la Camera dei Deputati ha recentemente approvato in modo *bipartisan* il disegno di legge sul cosiddetto controesodo. Si tratta in realtà della versione italiana della cosiddetta legge Beckham, adottata già diversi anni fa con successo dalla Spagna. È un primo passo e c'è da augurarsi che anche il Senato possa presto approvare tale provvedimento, ma non è certamente sufficiente. Un Governo, eletto anche col concorso dalla maggior parte degli italiani residenti all'estero che mi onoro di rappresentare, che si impegna efficacemente per la tenuta del sistema Italia e che è chiamato dagli italiani a riformare il Paese, non può, secondo noi, ulteriormente sottovalutare questa emergenza.

a un Esecutivo propenso ad alimentare i brillanti riti e a suonare il piffero delle magnifiche sorti e progressive, non certo abituato e peraltro poco credibile quando si rivolge al Paese per chiedere sacrifici. Non è abituato, perché questo Governo non ha mai dismesso gli abiti gattopardeschi: cambiare tutto perché nulla cambi. L'Esecutivo si muove consultando la bussola dei sondaggi e della comunicazione e accorre laddove vi sia il caso mediatico conclamato, come per esempio i rifiuti di Napoli, ma latita dove vi sia tale identica urgenza, come a Palermo. Siamo di fronte a una politica che rischia continuamente di redimere il falso e che, per converso, è autenticata solo dalle sue dichiarazioni. Sono sotto gli occhi di tutti la desolante trafila del caso Brancher, le riforme salva *Premier* o che nel migliore dei casi sono razionalizzazioni mascherate, volte solo al risparmio, effetti di una crisi troppo a lungo negata e rimossa. Sarebbe certo iniquo e ingeneroso cadere nella trappola che sempre si manifesta nella dialettica parlamentare degli schieramenti. Si è capito subito, fin dal suo affiorare, che una crisi di tale entità non è responsabilità di un Governo o di uno schieramento. I problemi, semmai, sono altri. Dovremmo capire, in particolare, che tipo di risposta si vuole fornire a delle domande che vanno ben oltre il momento contingente, ad una situazione che sul medio termine rischia di creare, come in parte è già accaduto, insicurezza, disparità sociale,

di don Paolo Gessaga, una povertà meno apparente ma più profonda, diffusa ed afona al pari della disuguaglianza. Molto ci sarebbe da dire anche sul sistema dell'informazione nel suo complesso, anche a prescindere dalla legge sulle intercettazioni. Nell'arco della stessa giornata, a commento dei più recenti dati ISTAT divulgati da ultimo, il TG1 annunciava la crescita del PIL come un timido accenno di ripresa, mentre il GR2 sottolineava un un picco della disoccupazione salito a sopra l'8 per cento, cosa che non si verificava da 30 anni a questa parte. Non solo: il 2011, da questo punto di vista, non promette nulla di buono; forse, le cose cominceranno a migliorare dal 2012. È senza lavoro un giovane su quattro ed un lavoratore su due ha un contratto cosiddetto atipico. Mi chiedo se questo sia lo stesso Paese in cui la voce del Presidente del Consiglio in una *spot* recentemente divulgato invita a trascorre le vacanze. Credo ci Credo ci si sia per troppo tempo nascosti dietro un sistema che, messo sotto pressione (è finita da un pezzo l'epoca delle vacche grasse), rischia di non credere più a quelle verità che stancamente ripete, perché è il sistema stesso che deve essere ripensato

sera e mattina - ha resistito meglio di altri alla crisi. Di quel Governo vediamo solo uno spogliatoio litigioso e un far melina inconcludente senza afferrare il nocciolo La Lega è disorientata dal vestire contemporaneamente i panni della forza di lotta e di governo; Fini e il suo gruppo scalpitano; governatori e industriali gettano il guanto di sfida, ma l'unica urgenza sembra quella di ridisegnare una legge sulle intercettazioni che, per la salvaguardia di pochi di pochissimi, ci fa tornare indietro di trent'anni, nel medioevo prossimo venturo. La vecchia favola dei ricchi sempre più ricchi che faranno star meglio anche i poveri emerge oggi nella sua evidente iniquità, nella sua storica inconsistenza.

Nel Paese delle frecce rosse e d'argento il biglietto più salato continuano a pagarlo i dipendenti pubblici, pendolari dei trenini locali. Ma forse il ministro Brunetta ci dirà che è giusto così perché sono fannulloni. Mi ha colpito, la scorsa settimana, Claudio Baglioni, ospite presso il premio Rodolfo Valentino, perorare, insieme con la causa di Telethon per la ricerca, l'equità e la dignità del pagare le tasse, vera e unica forma di giustizia sociale. Mi ha colpito perché un'affermazione così innocua è suonata, nella distratta e morbida quiescenza del piccolo schermo, come qualcosa di eversivo, di rivoluzionario. La Nazionale - scriveva Ilvo Diamanti dopo il crollo subito ai Mondiali - non è lo specchio della Nazione e neppure del Paese; è uno specchio di comodo, appunto, in cui rispecchiarsi quando conviene, a seconda Una manovra così concepita assomiglia più forse - in un Paese come l'Italia, dove la gestione della mediocrità, sebbene negata e invisa, è divenuta suo malgrado uno sport nazionale sport nazionale - ai tentativi, modesti e insufficienti, di arginare la marea nera nel Golfo del Messico. Questo Governo sta offrendo risposte altrettanto inadeguate: senza un ripensamento della società nel suo complesso e senza il coraggio della volontà, fuori dalle logiche corporativistiche che fanno arenare qualunque qualunque vocazione riformistica, non si andrà lontani. Questo rimane un Paese a due velocità: tapperemo una falla oggi per vederne affiorare innumerevoli in un prossimo futuro, quando la lentezza e i ritardi di tanti piccoli treni si ripercuoteranno sulle più lunghe percorrenze cui sono legate fiducia e speranza nel domani.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche la discussione generale ha offerto ulteriori il fatto che la manovra è necessaria, che le sue dimensioni sono adeguate e che ciò mette l'Italia al riparo da turbolenze finanziarie che

di affrontare le sfide anche nel prossimo futuro. Questa manovra è stata il sigillo ed il coronamento

Guido Carli individuò come uno degli ostacoli più grandi per l'impresa italiana. Penso che siano stati posti dei presidi essenziali. Molto si potrà migliorare, ma certo la strada per la semplificazione amministrativa è aperta, è stata aperta anche con quelle zone «a burocrazia zero» che mi auguro possano esprimere tutto il loro potenziale. Vi è quell'apertura straordinaria sulla compensazione tra debiti e crediti della pubblica amministrazione, che è un provvedimento che si inserisce - come ho già detto - nella linea strutturale di un nuovo rapporto tra pubblica amministrazione e fornitori e, per altro verso, di vero e proprio ossigeno finanziario per le imprese, che in questo momento ne hanno bisogno. poi la riscoperta delle reti di impresa, ed altro. Credo quindi che alcune questioni siano state ben affrontate. Non mi dilungherò sul Mezzogiorno d'Italia: troppo si è detto e troppo si è polemizzato. Forse

ha potuto ingenerare qualche confusione, penso che il Governo possa tranquillamente metter mano a quella proposta e rimediarvi, facendolo però proprio con il rispetto che si deve al dibattito parlamentare. Poi ci sarà la solita polemica fuori, ma pazienza. Penso che

su *input* del Governo e con le orecchie sensibili alle parti sociali e alle altre istituzioni. Questo mi pare il segno di ciò che é avvenuto

dopo questa discussione, abbiamo svolto ancora il nostro buon lavoro. Colgo l'occasione, signor Presidente, per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa manovra; li ringrazio veramente di cuore e dico sempre: è stato un onore aver partecipato con loro alla stesura di questo di questo importantissimo provvedimento. credo che le argomentazioni che abbiamo ascoltato in Aula, dai banchi sia della maggioranza che dell'opposizione, confermino

molti interventi hanno sottolineato che questa manovra finanziaria in fondo è in linea con le manovre attuate in altri Paesi europei. Che cosa è mancato Che cosa è mancato al nostro Paese? È mancato che in questa manovra non vi è stato un benché minimo, timido accenno ad una giustizia redistributiva. In Gran Bretagna, presidente Azzollini, è stata approvata una manovra finanziaria in cui, tra l'altro, è stata introdotta la tassa sulle rendite finanziarie: noi dell'Italia dei Valori, nel nostro pacchetto di 150 emendamenti, avevamo proposto - riscontrando, lo devo dire, anche una certa ironia da parte della maggioranza - la tassazione sulle rendite finanziarie. In Germania hanno istituito la tassa sul nucleare per il mantenimento di 17 imprese che provvedono alla gestione delle centrali nucleari e stanno definendo nel dettaglio la tassa sulle banche;

Gli altri Paesi si stanno muovendo verso una direzione di giustizia redistributiva, la grande assente di questa manovra Signor Presidente, non dobbiamo commettere l'errore di dividerci tra i rigoristi, che credono che la stabilizzazione dei conti pubblici sia il primo ed esclusivo passaggio, e chi invece sostiene

l'inflazione, sulla quale non riusciamo ad agire; il tasso d'interesse sul debito, su cui non riusciamo ad agire; infine, il terzo fattore, il tasso di crescita. crescita. Se vogliamo veramente sostenere la credibilità del nostro debito sovrano, dobbiamo agire subito, non tra otto mesi, quando rifaremo un'altra nuova manovra correttiva. Dobbiamo agire subito su questo elemento del saldo primario, determinato dalla crescita del nostro Paese. Nel merito, Presidente, questa manovra finanziaria presenta un piccolo specchietto dell'immagine che stiamo offrendo al Paese.

delle indennità di due Ministri e sette Sottosegretari per un risultato complessivo di 72.000 euro. Questo è lo specchio che la manovra economica presenta al Paese. Paese. Presidente Azzollini, conosco l'inglese meno di lei. Però c'è un bel proverbio inglese che vorrei ricordarle: non si riesce a fare una frittata se non si rompono le uova. Questa è una frittata uscita male, e avete rotto le uova sbagliate. approfitto di questi cinque minuti per sollevare alla Presidenza anche un problema di organizzazione dei nostri lavori. Anche in questa occasione, come è prassi del Senato in presenza di un decreto-legge, non si prevede la pubblicazione di un testo Commissione del provvedimento. Dunque, noi abbiamo svolto tutta la discussione generale senza poter conoscere gli oltre 60 emendamenti approvati in Commissione se non attraverso una faticosissima ricerca

presentati. Vorrei quindi sollecitare la Presidenza a valutare la possibilità che, in occasione di decreti-legge

di materie tra loro molto differenziate, sia possibile prevedere la pubblicazione di un testo Commissione del provvedimento che consenta all'Assemblea di lavorare avendo una base conoscitiva certa del testo, su cui si agisce poi anche con emendamenti. Infatti, per formulare gli emendamenti ai provvedimenti usciti dalla Commissione dobbiamo usare lo strumento ovvio dei subemendamenti. Mi sembra che quando c'è una materia complessa si potrebbe prevedere,

voglio sollevare di fronte al relatore due questioni specifiche, perché dagli aspetti puntuali si vedono anche i difetti propri di un eccesso di pressappochismo, di superficialità di alcuni aspetti della manovra. In Commissione abbiamo fatto una battaglia politica molto dura sulla questione dell'invalidità. La proposta iniziale del Governo era inaccettabile: colpiva i veri invalidi, e non i falsi invalidi.

Non si capisce perché ancora una volta bisogna pervicacemente agire sui più deboli della società. Voglio cogliere l'apertura che il relatore ha fatto nella sua replica

Con un emendamento in Commissione è stata prevista l'abolizione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale

delle scuole primarie e dell'infanzia. Non gode di alcun contributo pubblico, non si occupa di previdenza, perché interviene nel campo assistenziale integrando l'assistenza di carattere medicale, i soggiorni estivi, ed ha un patrimonio proprio, costruito nel tempo attraverso i contributi degli associati. Cosa c'entra l'INPDAP, che è un ente di carattere previdenziale, ed il fatto che lo Stato si appropri

Rinnovo a lei, signor Presidente, e al Ministro la nostra proposta: siamo disponibili a ridurre a 25 i nostri emendamenti;

Se non ne volete discutere non è perché manca il tempo: non volete discuterne perché la vostra maggioranza è divisa sul giudizio sulla manovra. Non siete capaci di affrontare un confronto chiaro in Aula di fronte all'opinione pubblica, ma questo è un modo di impoverire la vita democratica del Paese.

poche considerazioni. La prima la rivolgo ai relatori di minoranza, e riguarda la cornice complessiva, che ha ovviamente valenza politica. Tutte le proposte delle opposizioni, per quanto interessanti e autorevoli, soprattutto in materia di sviluppo (la linea che è stata seguita è, da una parte, politiche di rigore della spesa, dall'altra, necessità di ulteriori "iniezioni" sullo sviluppo)

delle rendite finanziarie e a interventi, anche retroattivi, per quel che riguarda lo scudo fiscale. Queste norme prevedono un innalzamento della pressione fiscale come scelta politica, che noi ovviamente rispettiamo, nel dibattito maggioranza-opposizione. È giusto ribadire che il Governo ha fatto una scelta diversa, lavoriamo per modificare e ridurre la spesa pubblica, consolidando comunque le dinamiche di controllo della spesa e del debito, che che sono elementi fondamentali inseriti in un coordinamento di politiche finanziarie premiate ancora oggi e considerate anche in sede Ecofin come dati positivi che l'Italia porta all'Europa.

di assoluto rilievo ed hanno in maniera significativa cambiato il testo: un testo che è stato discusso per davvero in tutte le sue parti. il sottosegretario Casero abbiamo potuto evidenziare in queste dinamiche un'analisi approfondita. Credo sia questo un elemento di merito del Senato, che è riuscito sulle questioni prioritarie, ricordate correttamente nella relazione del presidente dare segnali importanti per avvicinare ulteriormente la sensibilità e la scelta del Governo in merito alla tenuta dei conti pubblici, e ovviamente del sistema Italia di fronte a questi rischi congiunturali e di crisi dei mercati,

In merito, senatore Giaretta, credo ci sarà ancora attenzione su alcuni temi posti dall'opposizione. Il Governo è comunque sensibile, mantenendo però una cornice di fondo: quella della tenuta

credo però che questo messaggio da parte del Governo sia importante per poter concludere al meglio, approfondendo, anche nelle prossime ore, il lavoro svolto, rispettando al massimo l'operato della Commissione.

a questo punto, considerato l'ampio confronto parlamentare che c'è stato in Commissione e in questi giorni in Aula, come è stato ricordato dal presidente Azzollini (e volevo unirmi anch'io alle parole di ringraziamento a tutti i commissari

78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, attesa la straordinaria importanza che il Governo attribuisce all'approvazione in tempi certi di questo provvedimento.